l'aumento della spesa corrente, la diminuzione delle entrate primarie e, quindi, complessivamente, una difficoltà dei nostri conti pubblici ha fatto emergere un forte disagio sociale, caratterizzato dalla comparsa e dall'aumento di nuove forme di povertà e anche dall'accentuarsi delle diseguaglianze tra i cittadini. Questo ha avuto dei riflessi anche in campo sanitario. Il nostro Paese dal punto di vista sanitario si è aperto al nuovo millennio presentando due dati. Il primo è un aumento del tasso d'invecchiamento della popolazione, il che dimostra come i servizi sanitari e il Sistema sanitario nazionale

l'ambito sanitario e sociale è il miglioramento complessivo, il progresso che si è avuto in questi ultimi decenni in campo medico e diagnostico a livello internazionale, ma anche grazie al contributo italiano. Il DPEF, preso atto di questi due macroelementi, individua e cerca d'intervenire su alcune criticità presenti nel nostro sistema, quali l'inappropriatezza di alcune prestazioni e la conseguente migrazione interna dei pazienti verso livelli di maggiore qualità di cure; si pensi alla migrazione dal Sud al Nord del Paese, ma anche all'interno di alcuni ambiti regionali, alle lunghe liste d'attesa, all'elevata spesa farmaceutica che riguarda in modo particolare alcune Regioni. Obiettivo del DPEF è quindi quello di massimizzare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, così da far sì che la sanità possa svolgere pienamente il suo ruolo sociale ed economico. La spesa sanitaria viene quindi definita - e questa è la prima affermazione di principio importante - come forma essenziale di investimento nel capitale umano e la sanità viene individuata come una delle priorità più importanti su cui investire. Uno dei primi atti compiuti da questo Governo è stato infatti un nuovo patto con le Regioni riguardante il sistema sanitario, al fine di far rientrare entro il 2009 il forte disavanzo che caratterizza in modo particolare alcune aree del Paese. A tale proposito, il DPEF individua un fondo straordinario, decrescente nel tempo, in grado di azzerare totalmente i disavanzi attraverso un doppio impegno: la corresponsabilità regionale, avvalendosi inizialmente della fiscalità generale. Complessivamente il DPEF offre due messaggi. Innanzitutto un messaggio rassicurante verso il cittadino paziente, colui che ha bisogno di cure, il quale viene rassicurato che i livelli essenziali in campo sanitario saranno garantiti. Il secondo messaggio è rivolto invece alle Regioni per una corresponsabilizzazione delle stesse. Credo che complessivamente questo capitolo del DPEF possa essere riassunto nella seguente affermazione: «garantire di più per garantire meglio», attraverso il binomio «autonomia e responsabilità». La spesa sanitaria dell'amministrazione pubblica nell'ultimo quinquennio, lo ha ricordato il relatore Morgando, è aumentata di un tasso medio del 4 per cento e l'incidenza sul PIL è passata dal 5,7 al 6,7 per cento; un *record* negativo, negativo, non solo perché la spesa sanitaria è aumentata, ma perché non è stato proporzionale l'aumento dei livelli essenziali di assistenza garantiti ai cittadini. Voglio citare alcune patologie. Si pensi, ad esempio, alle patologie rare (i pazienti che sono affetti sono stati isolati e abbandonati a loro stessi) o alle risorse finanziarie per il personale medico e paramedico (il rinnovo del contratto dei medici è stato fatto solo nel 2005, ed era scaduto nel 2000). Ci sono quindi elementi di fortissima criticità. Le Regioni devono conoscere le risorse disponibili a loro destinate in modo da poter programmare le politiche da attuare, il contenimento delle spese da effettuare e il riassorbimento delle eventuali inefficienze. Non solo: l'autonomia fiscale in caso di disavanzo comporterà una maggiore responsabilità e autonomia nella gestione patrimoniale. Il percorso da fare parte proprio da un atto di fiducia che trasforma il controllo fiscale in un'ipotesi progettuale che possa realizzare uno sviluppo equo e solidale del sistema sanitario nazionale, così da garantire servizi essenziali per i cittadini distribuiti su tutto il territorio nazionale. Chiedo ancora Chiedo ancora un minuto, e concludo, per individuare le priorità. Innanzitutto è stata individuata la priorità della non autosufficienza, soprattutto per gli anziani soli e lasciati a loro stessi. L'altra priorità su cui lavorare è quella dei medici di famiglia, che sono uno strumento importante per la prevenzione, e possono garantire attraverso i medici associati un servizio migliore per i cittadini. Infine, il DPEF individua la priorità dell'infanzia. La maternità e l'infanzia restano due priorità importanti. Credo quindi che questo Documento, senza essere un libro dei sogni,

i quali, peraltro, non sono né così puntuali né così certi. Il ministro Visco ci ha abituati a delle a delle papere in termini numerici abbastanza consistenti per potere prendere sul serio alcuni dati. Dico solo che, probabilmente, la manovra

del 1992 è qualcosa di pazzesco e inaccettabile, visto che stiamo parlando di 70.000 miliardi di vecchie lire e di una manovra di dimensioni mai replicate dopo quella data. Se solo consideriamo la capacità depressiva rispetto all'economia che tutte le manovre hanno avuto, possiamo ben capire che effetti avrà questo tipo di manovra.

collega Baldassarri, di inserire questo Documento programmatico in una visione geopolitica assolutamente in movimento e variabile, che non vede più alcuni Paesi industrializzati come trainanti dell'economia mondiale, basti pensare a ciò che sta accadendo con la Cina, con il Brasile e con l'India, per capire che questo Documento non è altro che la declinazione delle vaghezze del programma elettorale dell'Unione. A questo aggiungo anche gli aspetti all'Europa, i parametri di Maastricht e, soprattutto, il cambio euro-dollaro che sono stati gli elementi fondanti di una certa regressione economica e non hanno permesso uno sviluppo economico

che l'accesso al credito, l'internazionalizzazione e l'innovazione delle piccole e medie imprese si realizzano solo cercando di far fare «dimensione» a queste aziende ebbene non ho trovato un solo capitolo o un solo argomento

fare di questo comparto, che è ritenuto da tutti, Comunità europea compresa, l'unico grande vero elemento di sviluppo per i Paesi industrializzati nei prossimi dieci-vent'anni.

Signor Presidente, signor Ministro, credo non sia utile sottacere in questo dibattito che la discussione avviatasi sul DPEF all'indomani della sua approvazione da parte del Governo in evidenza che l'impianto della politica economica ha costituito, nelle scorse settimane, uno dei punti di criticità nel confronto interno alla maggioranza. Come è noto, il ministro Ferrero non ha votato in seno al Consiglio dei ministri il DPEF e problemi sono sorti nel rapporto tra il Governo e i sindacati. Ora, come anche la discussione sin qui svolta dimostra, siamo molto avanti rispetto a questo stato delle cose ed elementi di coesione si sono introdotti nel dibattito all'interno della maggioranza. Tuttavia, voglio dire che nelle scorse settimane ho condiviso molte delle contrarietà e perplessità emerse all'interno della maggioranza. Non sfugge, infatti, a nessuno che il fatto che si individuino nel sistema pensionistico, nella sanità, negli enti locali e nella pubblica amministrazione le fonti da cui trarre le risorse per il risanamento dei conti pubblici sottopone inevitabilmente ad una ulteriore pressione i capitoli principali su cui è costruita la nostra spesa sociale, già ampiamente ridimensionata dall'azione di governo della destra, che ha portato i nostri conti fuori controllo, soprattutto per la sciagurata politica delle entrate e per il mancato controllo della spesa corrente più che per una politica della spesa sociale, che non è stata nel quinquennio che abbiamo alle spalle particolarmente generosa. Vedremo con la legge finanziaria che cosa accadrà. Comprendo, naturalmente, che il Governo si è trovato di fronte ad una situazione dei conti pubblici ben più grave di quella a cui si pensasse al momento della elaborazione del programma dell'Unione. Il riferimento alle condizioni del 1992 è troppo forte per essere semplicemente di maniera, come sostiene l'opposizione, né mi sfugge quanto impegnativa, dal punto di vista finanziario, sia la realizzazione del principale obiettivo che abbiamo posto in campagna elettorale: mi riferisco a quella riduzione del carico fiscale e contributivo sul lavoro delle imprese - altro che aumento della pressione fiscale - nota come riduzione del cuneo fiscale. Apprezzo anche la correzione di rotta che il DPEF avvia sulle politiche del lavoro, del lavoro, rimettendo al centro delle politiche del Governo azioni di sostegno all'allargamento dell'occupazione e alla promozione del lavoro a tempo indeterminato, anche se non è ancora del tutto chiaro con quanta coerenza e compiutezza riusciremo poi a continuare lungo questa strada.

patto con le forze fondamentali del Paese, a partire dai sindacati dei lavoratori fino alle organizzazioni degli imprenditori. La risoluzione della maggioranza che voteremo alla fine di questo dibattito penso che incominci ad andare in questa direzione e spero che l'apertura di tale confronto caratterizzi il tempo che ci separa dalla legge finanziaria.

Toccherà al confronto che apriremo sulla finanziaria dover fugare questi timori che non sono solo miei ma dei sindacati e di tanta parte dei lavoratori. Per ultimo, vorrei è necessario dare un risalto maggiore nella risoluzione della maggioranza ai temi del Mezzogiorno e dare a essi la centralità strategica che avevano nel programma dell'Unione. La seconda questione è come si affronta la questione salariale e retributiva nel nostro Paese. Il DPEF fissa al 2 per cento il tasso di inflazione programmata. Ebbene, io ritengo che sarà difficilmente sostenibile, di fronte a un travaso di lungo periodo nella distribuzione del reddito nel nostro Paese

auguro che la nostra discussione nei prossimi mesi ne tenga conto, per mantenere quella coesione sociale di cui la maggioranza di centro‑sinistra ha bisogno.

intervengo per preannunciare il voto contrario al Documento di programmazione economico-finanziaria presentato dal Governo e per illustrare qualche riflessione, come già hanno fatto i miei colleghi di Alleanza nazionale. Il DPEF, così come prevede la legge istitutiva del 1978,

Noi abbiamo letto questo Documento e abbiamo notato, con nostra sorpresa, che esso non contiene alcuna indicazione forte di politica economica, non contiene alcun respiro riformatore, non affronta il grande problema infrastrutturale del Paese che il Governo Berlusconi invece ha cercato di affrontare con la legge obiettivo. Il Documento contiene, a nostro avviso, solo un approccio penalizzante nei confronti dei ceti produttivi per i quali si prospetta, ahimè, un futuro di lacrime e sangue dal punto di vista fiscale, come è stato illustrato dall'onorevole senatore, relatore di minoranza Baldassarri.

leggendolo, infatti, si capisce che voi avete cambiato idea nei confronti del Governo Berlusconi dopo appena tre mesi. Leggiamo infatti nella pagina di trasmissione dell'atto l'obiettivo è «sbloccare un vero e proprio intreccio perverso nel quale si è venuta a trovare l'economia italiana dopo avere accumulato, a partire dalla metà degli anni Novanta, un ritardo di crescita che ha accentuato sia l'instabilità macroeconomica sia il disagio sociale». Quindi, il disagio sociale e l'instabilità economica partono dal 1995 e, se ricordo bene, questo Paese lo avete governato voi dal 1995 al 2001, per sette anni. A pagina 19 c'è anche un altro richiamo,

Ancora a pagina 23, vi è il confronto con le previsioni del DPEF 2006-2009; è scritto: «le previsioni macroeconomiche correnti per il 2006 confermano sostanzialmente quelle elaborate nell'ambito del DPEF dello scorso anno». Quindi, non è vero - come da voi sostenuto - che la nostra era una legge finanziaria di tipo elettorale.

poi nel Documento un accenno all'equità; non si sa come volete combattere l'evasione fiscale, ne parlate da mesi, tutta la vostra politica economica, il risanamento dei conti pubblici parte dalla

dell'evasione fiscale: voi non conoscete gli evasori fiscali, voi non sapete in che realtà vivete! Vi invito ad immedesimarvi

L'evasione fiscale si combatte attraverso un rapporto di avvicinamento che ci deve essere tra il cittadino e l'istituzione: bisogna dare i servizi, ecco quello che noi oggi vi diciamo. L'obiettivo del Governo Prodi, secondo noi, è solo quello - come è stato annunciato più volte di demolire le grandi riforme strutturali che il Governo Berlusconi ha portato avanti con coraggio e con grossi sacrifici nel settore dell'ambiente, con la riforma della scuola e dell'università, della previdenza, della giustizia e del lavoro. Queste sono

Non è scritto, non è dato sapere se volete continuare a portare avanti il programma strategico delle grandi opere, se volete realizzare o meno la TAV in Val di Susa. Siamo fortemente preoccupati per quanto emerge dal Documento che oggi ci proponete.

prima pagina del Documento. Il programma che Prodi ha presentato in campagna elettorale faceva riferimento alla profezia credibile; il candidato *premier* sperava nel profeta, oggi si richiama ai filosofi e riporta una frase del grande filosofo Kant, cito testualmente: «Coloro che dicono che il mondo andrà sempre così come è andato finora...contribuiscono a far sì che l'oggetto della loro predizione si avveri». È un invito all'ottimismo, certo chi governa deve essere ottimista e a questo punto ricordo il pessimismo dell'allora minoranza,

ma siete sempre voi quelli che dall'opposizione, come dei menagrami, avete diffuso il pessimismo del «tutto va male»? concludere questo mio brevissimo intervento con un consiglio alla maggioranza, affinché si dia una regola di condotta, ispirata sempre alla verità delle cose e alla correttezza e voglio utilizzare un'altra citazione di Kant, che contiene un monito ad evitare le mistificazioni e a dire sempre la verità, cosa che non avete mai fatto.

Questa è la frase che ho trovato questa mattina: «Due cose mi occorrono per essere felice: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me». Dite al Presidente di far buon uso anche di questa citazione, non solo dell'ottimismo cui faceva riferimento la frase di Kant che ho citato prima, anzi vi invito a mettere in pratica entrambe le citazioni, se ci riuscite.

una legge dello Stato, la legge obiettivo, impone che alla presentazione del DPEF sia allegato un documento molto importante, l'allegato alle infrastrutture, che è appunto previsto sia dalla legge obiettivo, sia dalla legge n. Nell'allegato alle infrastrutture avrebbe dovuto essere approvato dal Governo, rispettando una chiara procedura, una sorte di liturgia, prevista appunto dalle leggi di riferimento, un documento in grado di indicare non solo delle analisi teoriche, non solo delle linee strategiche e degli approfondimenti fatti da uffici e studi all'uopo preposti, ma capace di definire quali saranno i precisi interventi concordati con le Regioni e supportati da un piano finanziario adeguato e quindi dimensionato nel breve e medio termine. Tutto ciò, signor Ministro, purtroppo manca.

di questa mancanza da noi considerata molto grave. Il Governo, punto nel vivo, ha cercato di correre ai ripari e, in particolare il ministro Di Pietro, si è impegnato in due occasioni, sia in Commissione che nel corso dell'annuale assemblea dei costruttori,

ufficio stampa del Governo Prodi, si è trovato costretto a dichiarare che il Governo non è in grado oggi di individuare le priorità per la realizzazione delleinfrastrutture, anche perché la situazione dei conti pubblici è difficile e non c'è chiarezza sulle risorse esistenti.

Di Pietro. Mi sembra una dichiarazione importante. Ricordo infatti che in campagna elettorale la disputa polemica tra la maggioranza uscente e l'opposizione di allora verteva sul fatto che secondo l'opposizione noi avevamo ingannato l'opinione pubblica, proposto opere pie, promesso

firmato da un Governo che nei suoi rappresentanti più autorevoli ha brillato per condurre una campagna elettorale ad alzo zero contro ciò che era stato fatto a livello infrastrutturale dal Governo Berlusconi e dal ministro

Qui si dice che avremmo illuso l'opinione pubblica, gli Enti locali, le Regioni perché abbiamo promesso cose che non siamo stati in grado di mantenere.

acquisito che abbiamo ricevuto in eredità un Paese nel quale non esisteva un parco-progetti anzi, il bagaglio progettuale non superava il 10 per cento delle opere che si potevano e voglio chiarire che anche nella rivisitazione compiuta dal CIPE soltanto sei mesi fa in ordine ai maggiori costi che si dovevano affrontare per realizzare le opere previste dal Piano decennale, questa soglia dei costi immaginati saliva a 173 miliardi.

Perché dico tre e non cinque anni? Anche questo deve essere chiaro. Abbiamo preso la gestione, la responsabilità del Governo nel maggio 2001. La legge obiettivo è nata alla fine del 2001; la delibera CIPE è del 21 dicembre 2001; segue la fondamentale, perché è la prima riforma organica e strutturale della legge Merloni che - ricordiamolo - ha paralizzato l'attività nel settore pubblico dal 1993 al 2001 in Italia, e siamo partiti operativamente alla fine del 2002. Quindi, abbiamo reperito queste

la religione delle risorse pubbliche. Le risorse pubbliche sono quelle che sono! Da Maastricht, dal 31 dicembre 1992, le risorse pubbliche sono sempre le stesse. Ciò che voi non capite, perché è lontano

hanno costituito in questi mesi il fondo-clessidra? Perché la Cassa depositi e prestiti fa un fondo chiuso per le infrastrutture, coinvolgendo privati? Perché i privati già oggi sono disposti a realizzare opere pubbliche perché trovano convenienza

tradizionale, superato di vedere le cose nel nostro Paese, signor Presidente. L'ultima riflessione è l'accusa di aver fatto una serie di opere, senza una logica programmatoria: abbiamo fatto ciò che ci

che sembra più scritto da studenti della scuola media superiore che non da gente che conosce la realtà nel nostro Paese. Prima di operare scelte, bisogna conoscere la domanda di infrastrutture e i livelli di prestazione funzionale, la distribuzione dei costi

rappresentiamo la nostra delusione ed il nostro rammarico che anche sulle cose vere, dimostrate *per tabulas*, ci sia da parte vostra questa insensibilità e questo non riconoscimento.

discutiamo oggi il Documento di programmazione economico‑finanziaria, cioè la scelta del Governo per i prossimi cinque anni del Paese (anzi, per il medio periodo), consapevoli che questo è solo l'inizio, ma che già da ora si intravede la strada. La scelta - com'è stato ampiamente detto - è su tre fronti, tra loro strettamente legati. Ma è una scelta unica, qui sta la novità politica: la crescita per generare risorse e, insieme, l'equilibrio di bilancio per una finanza pubblica sana, per ridare fiducia nell'investimento e sul futuro, e, insieme, l'equità sociale e fiscale. Di fronte a queste dichiarazioni bisogna soltanto dire che dobbiamo riuscirci, perché ne va della capacità dell'Italia di stare al mondo. È una scelta coraggiosa per dare speranza al nostro Paese, per farlo uscire dalla combinazione pericolosa

bloccate nelle loro possibilità (senza opportunità di lavoro e di vita), e di un impegno vero per combattere la povertà e l'emarginazione. Cioè - potremmo dire - non siamo rassegnati alla situazione grave del Paese; qui c'è una strategia per ripartire. Dico subito che il motore della crescita è la conoscenza. Prendo sul serio il fatto che il DPEF sceglie di assumere la strategia di Lisbona; la 7a Commissione del Senato, di cui faccio parte, ne ha ampiamente trattato. La conoscenza per la crescita: come si devono aprire i mercati, così si deve aprire ed ampliare la quantità e la qualità dell'istruzione, per tutte le età e le aree del Paese, per la nuova sfida dell'immigrazione. Ciò ha che fare con la ragione sociale europea,

C'è più che mai bisogno di questo sogno europeo e che in questo sogno ci stia l'Italia. Nel Documento del Governo la strategia per l'istruzione è chiara, ma intendo ribadirla in questa sede con grande decisione. Essa ‑ si dice ‑ verrà assicurata sin dai primi livelli del processo educativo, a partire dagli asili nido, potenziando il diritto allo studio attraverso l'estensione dell'obbligo scolastico, il potenziamento delle autonomie scolastiche, la messa a norma del patrimonio edilizio e l'incentivo all'utilizzo pomeridiano degli edifici. Non meno rilevante, in questo contesto, è la necessità di affrontare un problema cronico della scuola, il problema dei precari, nel quadro di un più generale programma di rimotivazione e di recupero della fiducia dei docenti e delle famiglie, oltre che di stabilità del sistema. Abbiamo un problema da risolvere nei prossimi anni: come colmare il divario con gli altri paesi nella comparazione internazionale sull'istruzione e come consentire a tutti i ragazzi del nostro Paese, non uno escluso, di inserirsi, con un'adeguata preparazione, nei continui mutamenti sociali, culturali, tecnologici dell'economia e del lavoro. E così è per l'università; vogliamo renderla più competitiva attraverso una gestione che premi il merito e la ricerca della qualità. Un passaggio decisivo per la crescita è dunque l'investimento in ricerca, la collaborazione tra imprese, università, centri di ricerca, anche attraverso il credito di imposta automatico, e la promozione di processi innovativi per un nuovo modello di politica industriale che sarà articolata per obiettivi e per progetti integrati locali, così da promuovere la competitività delle filiere produttive. Considero decisiva la strategia per il Mezzogiorno, come strategia dell'intero Paese: lì dovremo promuovere i talenti, le imprese, l'iniziativa, la cultura; la cultura perché i beni e le attività culturali strettamente connessi al turismo sono una ricchezza per l'Italia e lo sono per il Mezzogiorno. Lì è l'Europa nel Mediterraneo e sono parte di quel marchio Italia nel mondo che si intende rilanciare. Cultura e turismo, dunque, per fare dell'Italia ciò che deve essere nel mondo. In questo contesto, particolarmente significativa è la promozione dei cammini d'Europa, per noi la via Francigena, e degli itinerari storico-culturali e religiosi che sono a fondamento dell'unione politica dell'Europa. Sottolineo, infine, la necessità prevista di rifinanziare il Fondo unico per lo spettacolo, poiché grande è la creatività e straordinaria la capacità di produzione di spettacolo del Paese; è una ricchezza e un investimento nelle professioni dello spettacolo, è un investimento nell'economia oltre che nella cultura. Ecco dunque la forza dell'Italia: la scuola, l'università, la ricerca, la cultura, i beni artistici e culturali, il turismo e la capacità di iniziativa, di impresa, di innovazione. Soprattutto dei giovani e delle donne, che sono la grande potenzialità dell'Italia. Ci sono quindi le condizioni perché l'Italia ce la possa fare; ci vuole dunque il coraggio di scegliere, di decidere, di intervenire e non c'è tempo da perdere. Perché questo DPEF e la prossima finanziaria comincino a cambiare davvero la vita degli italiani e diano nuovo slancio al sistema Italia, come del resto è nelle attese del popolo italiano che, per parte sua, ha dato, con le elezioni, un nuovo Governo al Paese. Lo ha dato perché ci sia una nuova speranza per tutti.

Presidente, care colleghe e cari colleghi, i pochi minuti che mi sono stati assegnati e la complessità del Documento che stiamo discutendo mi costringono a fare due scelte molto secche su temi che mi stanno particolarmente a cuore, anche perché tutti gli altri sono già stati ampiamente trattati da colleghi con competenza e con puntualità. Il primo argomento che vorrei trattare è quello delle politiche territoriali, relegate alle ultimissime pagine del Documento, e in particolare la specificità delle zone di montagna. Il secondo tema è il turismo, inserito quasi come un corpo estraneo, in un contesto troppo generico ed accostato ai beni culturali con un matrimonio decisamente forzato, senza grandi rapporti, diciamo, né d'amore né di interesse. Il titolo di base del DPEF si ispira alle strategie varate a Lisbona, quindi improntate alla crescita, al risanamento e all'equità. I tre obiettivi sembrano sintetizzare i bisogni essenziali proprio delle zone di montagna, che sono totalmente assenti nelle 160 pagine del Documento di base e assenti anche nelle 233 pagine dell'allegato tecnico. L'Italia - tutti lo sappiamo - è un Paese prevalentemente montuoso: oltre il 70 per cento del suo territorio è costituito da montagne e da colline. Il 54 per cento dei comuni viene riconosciuto dall'UNCEM come comuni montani. Su questo territorio, però, vive soltanto il 15 per cento dei cittadini italiani, quindi una lobby piuttosto debole, a favore di questa specificità. Quando si parla di montagna non mancano - almeno a parole - molti sostenitori; forse per romanticismo, bontà d'animo, per consuetudine ma anche in questa legislatura, per esempio, è stato rilanciato il Gruppo interparlamentare "Amici della montagna" che conta a tutt'oggi poco meno di 200 tra senatori e deputati. Ci sono anche molti membri del Governo - non so se vi sia il vice ministro Visco - ma peccato che nel DPEF non si trovi

Vi hanno contribuito la risoluzione del 1998 sulle nuove strategie per la montagna in Europa, l'Anno internazionale della montagna del 2002 e l'azione convinta del Governo della Casa delle Libertà, che ha compiuto alcuni importanti passi per dare alla montagna dignità e il riconoscimento che merita. Innanzitutto, ha portato a termine l'impresa storica d'inserire nel testo della Costituzione europea, al terzo capitolo, il riconoscimento esplicito delle zone di montagna come una specificità da tutelare, insieme a quelle delle zone insulari e delle zone costiere; poi, ha istituito la giornata internazionale della montagna, d'intesa con le Nazioni Unite, fissandola per ogni 11 dicembre. Ancora, ha assegnato competenze - parlo sempre del Governo

Particolarmente importante è l'inserimento della specificità della montagna nel testo della Costituzione europea, ottenuto dopo un *pressing* formidabile sugli altri Paesi a conclusione del semestre italiano di Presidenza dal giugno al dicembre 2003. Al di là dell'aspetto politico e della soddisfazione politica, questo successo dischiude la strada a possibili iniziative molto concrete, ad esempio all'assegnazione di incentivi anche in deroga al regime degli aiuti di Stato, che divengono più elastici proprio in virtù dell'assegnazione della specificità nel testo costituzionale. Certo che, se a fronte di questa conquista i Governi - il nostro, per esempio - non rispondono con la dovuta attenzione, al danno, davvero, si unisce anche la beffa, ripensando alla fatica fatta anche in sede di Parlamento europeo per fare digerire la montagna a Paesi che proprio non ne volevano sapere. Nell'Unione Europea, infatti, la *lobby* della montagna è ancora più debole rispetto all'Italia: comprende il 40 per cento del territorio e Per questo considero doppiamente criticabile la mancanza nel DPEF di qualsiasi previsione a favore della montagna e a sostegno del ruolo importante che in queste politiche esercitano le Regioni, le comunità di valle e i Comuni. Questa amara constatazione non incoraggia certo coloro che stanno cercando di rilanciare la proposta di riforma della legge n. 97 del 1994 in attesa di aggiornamento ma, soprattutto, di una dignitosa dotazione finanziaria per essere reinventata. modo, occorre mettere mano con decisione al Fondo nazionale per la montagna perché non sia più una nicchia, qualcosa molto simile a un'elemosina. Eppure, nel DPEF si parla di esigenze di garantire a tutti i cittadini, in particolare ai giovani, alle donne e agli anziani, testualmente: «una maggiore equità per contrastare nuove forme di emarginazione sociale, di diseguaglianza e povertà». In montagna l'emarginazione è più lacerante che nelle altre località, la disuguaglianza è più desolante e, se così si può dire, anche la povertà è più povera. Pensate alla montagna, signori del Governo, quando al quarto capitolo parlate di dinamiche della produttività e dell'occupazione, oppure quando dedicate un inciso ai giovani, ricordando il Patto europeo per la gioventù, siglato l'anno scorso dal Consiglio per migliorare la loro istruzione, la formazione, la mobilità, l'inserimento professionale e sociale. Pensate a tutto questo applicato, per esempio, al figlio del montanaro che nasce in una malga del Trentino o della Valle d'Aosta o a qualche giovane agricoltore delle montagne più periferiche dell'Appennino. Pensate anche alle donne di montagna quando riaffermate il giusto diritto della donna, leggo testualmente dal DPEF, di «ampliare il diritto per le donne di partecipare al mercato del lavoro senza rinunciare al loro diritto alla maternità». Oppure al paragrafo dedicato alla famiglia si dice: «contrastare la povertà e l'esclusione sociale, con particolare riguardo alle problematiche della famiglia». Pensate sempre alle famiglie che vivono nelle zone più disagiate della montagna e al modo di applicare tutto questo anche lassù, perché anche lassù vi sono cittadini italiani. E ancora, per la parte riservata agli anziani, se la situazione non fosse drammatica, ci sarebbe persino un pochino da sorridere: di «(...) favorire una vecchiaia attiva, inserita nella rete delle relazioni affettive, familiari e sociali, assicurando nel contempo assistenza a chi ne ha bisogno». vecchiaia attiva, signor Ministro, in montagna spesso è inevitabile, se si vuole continuare ad invecchiare, nel senso di sopravvivere. E un forte pensiero alle zone di montagna vi invito a rivolgerlo, in riferimento ai capitoli che il DPEF dedica alle prospettive di potenziamenti dei servizi di base: gas, energia elettrica, telecomunicazioni, scuole, ospedali, trasporti, negozi di prossimità e così via. Anche tutto ciò deve arrivare fino nelle zone più lontane.

dell'attività a sostegno dei beni culturali. Per noi, il rapporto deve essere invertito: i beni culturali debbono servire per attirare turisti e recuperare il *gap* che l'Italia ha oggi nei confronti di molti Paesi europei e mondiali, e quindi a favore delle attività produttive

guarderà ai tempi degli interventi in maniera molto restrittiva perché altrimenti non riusciremo ad arrivare alla fine del dibattito se non a notte inoltrata.

Purtroppo, ancora una volta vediamo che il Mezzogiorno cumula una serie di primati negativi: la povertà, l'impoverimento dei ceti medi, la disoccupazione, in specie femminile e giovanile, l'insicurezza, la presenza della criminalità organizzata, sia nei settori di tradizionale attività, sia in quelli più «moderni», come la lucrosa gestione dell'immigrazione clandestina e della permanenza illegale nel nostro Paese. E vediamo una forbice che di nuovo si allarga tra Nord e Sud. Voglio che resti agli atti la mia preoccupazione, perché il centro-sinistra in campagna elettorale ha giustamente prospettato una terapia d'urto per il Mezzogiorno, che è stato assunto come scommessa di tutto il Paese: ricordo manifestazioni in cui ho sentito autorevoli posizioni, nel senso che «il Paese non crescerà, se non attraverso la crescita del Mezzogiorno». Vi è stata una campagna elettorale in cui il Sud ha avuto una sua centralità: è stato visto come punta avanzata del contatto con i mercati emergenti e con la forza economica crescente delle tigri asiatiche, con proposte sulla infrastrutturazione, sul sistema portuale, sulle autostrade del mare e così via. Ma oggi tutto questo va in un orizzonte molto lontano, molto fumoso. Capisco che da un DPEF non ci si possa attendere troppo, ma mi sembra che veramente siano insufficienti l'attenzione e il dettaglio di questa proposta,

Il Mezzogiorno ha condizionato la vittoria nel 2001 e nel 2006. Ora, se non riusciamo a dare risposta al Mezzogiorno,

per la sua solidità e per la solidità della coalizione. Stranamente il Sud, che è stato centrale per la vittoria nella competizione politica, è in una condizione di nanismo politico. Tale contraddizione sì traduce

ha allertato e allarmato il Governo e il Ministro qui presente sulla poca attenzione posta al problema del Mezzogiorno. Anch'io, che sono del centro-destra e della Casa delle libertà, ho avuto modo nei cinque anni passati di allertare il mio Governo

del «contratto con gli italiani», come anche altri colleghi della mia parte politica hanno voluto sottolineare, per quanto riguarda le grandi infrastrutture. Certo, è avvenuto anche, ed è il caso di ricordarlo, che durante una legislatura caratterizzata da un tasso di crescita molto basso, pari allo 0,6 per cento, a causa di una congettura

anche senza la minimanovra. Noi sappiamo perché si è voluta fare la mini manovra. Sulla base di queste premesse, con la mini manovra si è aumentata la pressione fiscale, caro Ministro, mascherandola come lotta all'elusione, provvedendo all'istituzione di una sorta di Grande fratello fiscale. Noi saremo attenti e vigili a che questo non accada se non nel rispetto assoluto delle prerogative dell'Italia e della sua libertà. È innegabile, egregio Ministro, signori rappresentanti del Governo, signor Presidente, che ciò deve determinare degli effetti negativi. Passando poi all'esame del quadro macroeconomico, vi è da dire che, a fronte dei segnali di ripresa che certamente sono riconducibili agli effetti strutturali e di medio periodo delle riforme attuate dal Governo Berlusconi, esistono anche alcuni fattori di rischio che il DPEF all'esame non considera in assoluto, *in primis*

per intervenire sull'aumento della bolletta energetica. Allo stesso tempo, il DPEF non considera gli elementi in base ai quali il tasso di crescita del PIL è stato rivisto in rialzo dell'1,5 per cento rispetto al 3 per cento. E ancora, sul piano macroeconomico, quello che più ci affligge ci preoccupa - ed è riportato proprio in un rigo della relazione - è se nelle previsioni di crescita il Governo abbia tenuto conto dei potenziali effetti depressivi sull'economia legati all'andamento del rapporto del cambio euro‑dollaro. È assolutamente inimmaginabile

*(FI)*. Esprimo un'ultima perplessità: altro che crescita, equità e risanamento finanziario. Con questa manovra si è cercato di proteggere la grande finanza, non soltanto quella statale ma anche quella privata, e si è posta poca attenzione, come diceva il collega Villone, al problema del Mezzogiorno.

ha dimostrato che se si avviano per davvero le liberalizzazioni, quelle serie e non quelle punitive, effettivamente questo Paese potrà riprendersi.

desidero innanzitutto ringraziarvi per la calda accoglienza che avete riservato a noi parlamentari eletti nelle circoscrizioni estere. Dopo gli eventi nazionali e internazionali dalle elezioni politiche ad oggi - particolarmente quelli delle ultime settimane - vi confesso che le ragioni che mi hanno portato a candidarmi si sono rafforzate nella mia determinazione per il raggiungimento degli obiettivi che ho posto alla base del mio programma elettorale. Permettetemi di enunciare alcuni di questi obiettivi, non in ordine prioritario, che pongo all'attenzione di questa Assemblea, affinché possano trovare adeguati e urgenti finanziamenti: potenziamento dei fondi e dei servizi consolari degli istituti di cultura e degli enti assistenziali; incremento dei programmi culturali italiani presentati attraverso gli istituti di cultura e facilitazioni alla comunità per accedervi; superamento delle drammatiche carenze negli uffici pubblici locali e nazionali e nei dipartimenti ministeriali responsabili dell'erogazione dei servizi agli italiani residenti all'estero; potenziamento dei finanziamenti ai programmi italiani nelle scuole elementari, medie e superiori e alle associazioni senza fini di lucro che li offrono; finanziamenti adeguati per la stampa e i *media* in lingua italiana; incremento dei finanziamenti per scambi culturali a tutti i livelli; incremento dei finanziamenti per borse di studio per studenti delle scuole medie, superiori e universitari e programmi di collaborazione tra università e aziende private per *staging* e formazione facilitazioni delle normative e delle legislazioni per scambi commerciali, economici e finanziari e potenziamento del sistema camerale all'estero; riforma della legge per il riacquisto della cittadinanza italiana; riforma dei COMITES e del Consiglio generale degli italiani all'estero; riforma, riqualificazione e rilancio di RAI International, secondo le linee strategiche proposte dal vice ministro Franco Danieli nella sua relazione alla Commissione affari esteri del Senato

esteri, cui hanno partecipato il ministro Gentiloni e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Levi; assistenza economica alle piccole e medie imprese di italiani residenti all'estero che importano e vendono prodotti del *made in Italy*; aggiornamento delle liste dell'AIRE e revisione del regolamento per il voto degli italiani all'estero; incremento dei programmi per il recupero al sistema Italia di quegli italiani che si sono affermati all'estero nei diversi settori produttivi e culturali finanziamento di programmi per il rafforzamento delle tradizioni territoriali e culturali che abbiamo fatto vivere anche nei Paesi di accoglienza. Onorevoli colleghi, è stato detto e scritto molto sul valore economico che gli italiani all'estero significano per il bilancio dello Stato italiano: rimesse monetarie, consumo dei prodotti *made in Italy*, divulgazione nel mondo delle nostre tradizioni e della nostra cultura che divengono ripetitori efficientissimi a propagare un'attenzione verso l'Italia che stimola il mondo a osservarci, a imitarci, a visitarci, ad apprezzarci e anche ad amarci e, di conseguenza, a portare risorse e introiti nelle casse del sistema Italia. Tutto ciò deve essere messo a regime. Intendo dire che noi italiani residenti all'estero dobbiamo essere considerati una risorsa permanente dell'Italia, non un'anomalia occasionalmente visibile e utilizzata. L'anomalia della mancanza di rappresentanza è stata corretta con il voto per corrispondenza e la creazione delle circoscrizioni estere, ma non è pensabile che si possano esercitare le funzioni della nostra responsabilità di rappresentanti parlamentari senza che ci vengano date le dovute risorse finanziarie per gestire tali responsabilità. Dobbiamo avere la possibilità di essere presenti

Nessun Paese moderno può progredire senza confrontarsi con il mercato internazionale, a partire dalla sua capacità di innovazione e di fare sistema. Le nostre comunità all'estero sono parte fondamentale di questo sistema ed è in esse che si individuano capacità

ci mettano nelle condizioni di poterlo fare al meglio. Ciò che chiediamo è una giusta attenzione alla messa a punto del nostro motore rappresentativo. PRESIDENTE. Le chiedo scusa,

Signor Presidente, si è sempre detto che il DPEF non è che un libro dei sogni. Ebbene, quando ho letto questo DPEF la prima riflessione è stata che mi sarebbe piaciuto che la maggioranza politica di cui facciamo parte avesse osato sognare di più. Avremmo voluto un DPEF che desse maggiori segni di discontinuità rispetto alla politica economica e sociale dei Governi di centro-destra e anche ai precedenti di Governi centro-sinistra, di cui Rifondazione Comunista non ha mai fatto organicamente parte. Ora che abbiamo un patto di legislatura con l'Unione, che abbiamo insieme stilato un programma di Governo nel quale le istanze sociali hanno trovato ampio spazio e sul quale il popolo italiano ci ha dato fiducia, permettendoci di governare, avremmo voluto qualcosa di più. Ed è per questa, diciamo, timidezza del DPEF che il ministro Ferrero ha voluto segnalare il proprio disagio nella compagine ministeriale non partecipando al voto. Infatti, ci preoccupa fortemente la prospettiva di tagli alle spese sociali che intravediamo in controluce nel DPEF. Questo DPEF, infatti, fa sicuramente significativi passi avanti rispetto al quadro di riferimento della politica economica che questo Governo intende portare avanti rispetto all'impostazione del passato. Ma forse non li fa altrettanto nella concreta definizione delle misure da adottare per arrivare davvero a una nuova politica economica e finanziaria che abbandoni le politiche neoliberiste che hanno acuito enormemente privilegi e ingiustizie, rendendo sempre più ricchi i ricchi e spingendo addirittura sotto la soglia di povertà milioni di cittadini, e in particolare di cittadine (perché nel nostro Paese la povertà è sempre più donna) non solo appartenenti a fasce marginali, ma anche alla classe lavoratrice e alla classe media, che, in una società ormai caratterizzata dalla precarietà e da una corsa al rialzo dei prezzi senza freni (si pensi, prima fra tutti al problema della casa), vengono sempre più sospinte verso il basso. Serve, perciò, un'inversione netta verso un modello di sviluppo sostenibile ed equo, senza cedere e farsi adescare, come invece sembra avvenire in alcune parti, dalle sirene del neoliberismo, fondato sul mercato, sulla competitività, sulle privatizzazioni, su un'idea di sviluppo da cui è assente l'equità. Alcuni enunciati ci sembrano troppo vaghi, soprattutto per quello che riguarda il piano sociale. Il nostro impegno e la nostra lealtà verso questa maggioranza si concretizzeranno nel fare in modo che agli impegni seguano nella prossima finanziaria scelte concrete, per il diritto alla casa, per la rete degli asili nido, per la sanità, l'occupazione, le reali pari opportunità per le donne, in particolare nel lavoro e nella «conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro», che però riguarda tutti, non solo le donne. Per questo Rifondazione Comunista ha lavorato affinché la risoluzione proposta dalla maggioranza impegni il Governo a mettere in campo un'economia con una cifra del tutto diversa, un'economia che valorizzi invece di umiliarle le risorse umane, che si basi sulla lotta all'esclusione, che rispetti, invece che devastarli, i territori e il patrimonio ambientale, che sostituisca a una competitività senza regole la cooperazione economica e sociale, che tuteli con mezzi concreti, e non solo sbandierando principi che poi rimangono vuoti, l'uguaglianza economica e sociale di tutti i cittadini, i diritti sociali, l'equità, le pari opportunità, l'inclusione delle categorie svantaggiate, prima tra tutti quella degli immigrati, garantendo l'accessibilità ai servizi. Una risoluzione che impegna il Governo a evitare che il risanamento dei conti pubblici passi ancora una volta dal taglio della spesa pubblica, dall'attacco alle pensioni, alla sanità, agli enti locali. Il risanamento deve concentrarsi, e sarebbe veramente la prima volta, sulla lotta all'evasione fiscale, ma anche, com'era nel nostro programma, sulla tassazione delle rendite finanziarie, sul ripristino della tassa di successione sui grandi patrimoni, garantendo il principio costituzionale della progressività dell'imposizione fiscale. Per quanto riguarda la questione sociale, non vorremmo quindi che il DPEF finisse per condizionare l'erogazione dei servizi ai cittadini ai vincoli di bilancio; per questo riteniamo estremamente positiva la previsione di un potenziamento del fondo per le politiche sociali e la scelta, accanto al piano straordinario per la costruzione di 3.000 asili nido (perché di servizi hanno bisogno sopratutto i bambini e i genitori), dell'assegno per i minori; vorrei definirlo un reddito di cittadinanza del bambino, un reddito minimo d'inserimento che pone al centro la soggettività di ogni bambino e di ogni bambina, riconoscendone il diritto soggettivo, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali del nucleo famigliare in cui si trova a nascere e a crescere, a un'infanzia non tarpata dalla povertà, con tutte le conseguenze che questo può avere sullo sviluppo della persona e sull'inclusione sociale. Colgo l'occasione, anche se fuori tema, per fare un plauso all'attuale Governo per aver scelto di sanare una piccola ma significativa ferita vergognosa lasciata in eredità dal precedente Governo: avere abbandonato quel braccio di ferro con quei genitori che, avendo l'unica colpa di aver dato credito alla lettera ricevuta direttamente dall'allora Presidente del Consiglio, avevano riscosso il *bonus* *bebè*, una misura demagogica ed elettoralistica che pure noi non condividiamo, ma che non potevamo accettare divenisse ulteriore fonte di discriminazioni. Ancora, abbiamo ritenuto indispensabile prevedere nella risoluzione la stabilizzazione della spesa sanitaria (ricordo che ancora oggi è inferiore alla media europea), la stabilizzazione rispetto al PIL agli attuali livelli (6,8 per cento) attraverso una piena responsabilizzazione delle Regioni, in modo da garantire a tutti i cittadini livelli essenziali d'assistenza, ma credo che sarà anche necessario ripensare a come questa spesa si forma, ricordando che tutti gli studi internazionali ci dimostrano che un servizio sanitario fondato sul privato costa di più ed è meno efficace rispetto ad un servizio pubblico e che quindi la spesa va controllata non tanto a partire dalla spesa corrente quotidiana, ma sul piano strutturale. Abbiamo basato la nostra campagna elettorale su un messaggio centrale: legare politiche di sviluppo compatibili con una politica sociale basata sull'equità e l'equilibrio sociale. Per chi era abituato a lavorare sui DPEF presentati prima, in questo troviamo parole fortemente innovative: l'equità e la redistribuzione, ma soprattutto noi lavoreremo affinché queste parole, insieme ai cittadini, ai sindacati, alle associazioni di malati, agli utenti, nella prossima finanziaria divengano cifre.

di natura critica, sperando che il relatore le voglia accogliere e possano essere inserite nella risoluzione conclusiva. La prima osservazione è questa: ho una certa perplessità sulla modulazione degli interventi proposti nel DPEF.

allora dobbiamo aver presente che il nostro DPEF agisce in un momento in cui c'è una debole inversione di questa tendenza; siamo di fronte ad una debole ripresa dello sviluppo economico. È allora essenziale, a mio giudizio, non fare operazioni che deprimano questa tendenza; anzi bisogna, fare in modo che questa tendenza venga incoraggiata, che, come si dice, il vento gonfi le vele. Ecco quindi il problema: la legge finanziaria che questo DPEF individua per il 2007 - non tanto quindi la manovra quinquennale - rischia di avere un effetto in qualche modo depressivo. Individuo questo rischio principalmente in un elemento:

tra le risorse che vengono sottratte al prodotto interno lordo per la riduzione della spesa e le risorse che vengono iniettate.

l'effetto di riduzione complessiva della crescita per il 2007. Ebbene, poiché ritengo che questo effetto possa essere pericoloso, credo che sia giusto pensare ad una sua rimodulazione, cioè

considerando lo stato di realizzazione progressivo delle azioni strutturali che vengono compiute nella legge finanziaria del 2007, che potrebbero consentire di traguardare un periodo più lungo di tempo per la prima fase del rientro dal *deficit* del debito pubblico.

contro un'esigenza per la realizzazione di quel programma di investimenti pari a 111 miliardi di euro. Si è di fronte al reperimento del 18 per cento dei finanziamenti necessari al piano.

che aveva un piano di finanziamento di opere per 11 miliardi poi realizzato per meno di tre miliardi di euro, si ha l'immagine di quale sia lo stato effettivo dei lavori con i quali ci si deve confrontare. La terza osservazione riguarda il fatto che proprio per questa difficoltà e per questa grave insufficienza della realizzazione infrastrutturale in Italia, che è stata realizzata dal Governo di centro-destra, ci troviamo di fronte alla assoluta necessità di realizzare un piano straordinario di infrastrutturazione nel Mezzogiorno.

attualmente individuate per la realizzazione del Ponte sullo Stretto. Se il ponte non si farà, quelle risorse potranno servire al piano straordinario di opere infrastrutturali per il Mezzogiorno. *(Applausi

è stato costituito con grande strombazzamento il Ministero dell'ambiente e del mare: di pesca si parla solo per l'impatto ambientale, ma non si assegna al settore pesca, così importante nel nostro Paese (contiamo la prima flotta del Mediterraneo),

Pare che la lotta alla grande distribuzione organizzata del resto d'Europa, e in particolare francese, si possa fare solo e unicamente con la Lega delle cooperative. Quanto al cuneo fiscale, per fortuna il Governo Berlusconi ha abbattuto il costo del lavoro in agricoltura, considerato che il lavoro agricolo, come sa il ministro Visco, al 90 percento è costituito da lavoratori a tempo determinato. Con le opinioni del Governo attuale sul cuneo fiscale, il settore dell'agricoltura non avrebbe alcun beneficio. Concludo dicendo, caro Presidente, che il mio voto è tanto più contrario anche perché vedo che ancora una volta - è la seconda volta che la sinistra è al Governo da quando sono in Parlamento dopo le dichiarazioni svolte in campagna elettorale, cercando di richiamare i voti dell'elettorato agricolo e della pesca, da parte del Governo Prodi nei confronti dell'agricoltura, dell'agroalimentare e della pesca vi è uno zero assoluto.

Signor Presidente, nel mio intervento non citerò cifre o dati che già sono stati autorevolmente commentati da altri colleghi di maggioranza che mi hanno preceduto. Mi limiterò ad alcune osservazioni politiche che riflettono il mio sentire dopo la lettura e l'illustrazione del DPEF e la sua disamina in seno alla Commissione bilancio, alla quale ho partecipato. Del Documento ho innanzitutto apprezzato l'analisi precisa e per molti versi impietosa che, partendo da fonti ufficiali e diversificate, è venuta alla luce sulla reale situazione economica del nostro Paese dopo anni in cui i dati che venivano forniti erano a dir poco imprecisi e spesso sospetti di non essere del tutto veritieri. Mi sembra siano stati definiti opachi o oscuri dalla Corte dei conti. II lavoro di *due diligence* fatto dal Ministro ha ben evidenziato come i principali indicatori dell'economia nazionale (dalla bassa crescita alla produttività, alla quota italiana nel mercato mondiale, alla produzione industriale, al rapporto *deficit*-PIL per arrivare all'azzeramento dell'avanzo primario) siano andati costantemente peggiorando negli ultimi cinque anni e come siano in assoluto i peggiori anche all'interno dell'area euro, e quindi purificati delle pur presenti componenti congiunturali internazionali. È pur vero che segnali di preoccupazione si erano cominciati a vedere negli ultimi due anni di Governo del centro-sinistra precedente, ma non vi è dubbio che i cinque anni passati hanno segnato un netto peggioramento della nostra situazione e che in questi anni non si sono viste misure che intervenissero strutturalmente sui conti economici italiani, ma piuttosto ripetutamente misure *una tantum*, scarsamente efficaci sul piano economico e condannabili; mi riferisco, in particolare, alla politica dei condoni, sul piano dell'etica politica. L'accusa fatta più volte in Commissione e anche in Aula al Documento, cioè che vi sarebbe una sproporzione tra l'analisi tracciata e le misure adottate specie per l'anno in corso, non mi pare sinceramente fondata. Il DPEF traccia infatti un programma di legislatura con la giusta prudenza, che il ministro Padoa-Schioppa ha più volte richiamato nella sua presentazione. Programmare una crescita del PIL moderata ma costante è segno di saggezza, dopo le costanti sconfessioni di crescite brillanti programmate e poi sempre smentite, cui abbiamo dovuto assistere negli anni appena trascorsi. Realismo e prudenza, quindi, ben sapendo che, tanto quanto è difficile ritarare al ribasso le previsioni, adottando misure di contenimento sempre difficili e dolorose, altrettanto è piacevole per qualunque amministratore avere risorse aggiuntive da poter mettere in gioco nei settori più critici o bisognosi, quando queste dovessero generarsi. La suddivisione in tre fasi appare dunque ragionevole e ragionata, ma con un iniziale forte sforzo per rientrare al più presto nei parametri di Maastricht, secondo quanto ci chiede l'Unione Europea. La ripresa della produttività ed il miglioramento del gettito fiscale nel primo semestre di quest'anno sono sicuramente segnali incoraggianti, che in parte derivano da un miglioramento della congiuntura internazionale, ma certamente anche da un nuovo clima di fiducia che si è instaurato nel Paese con la vittoria del centro-sinistra e la credibilità del suo programma e dei suoi rappresentanti al Governo. Non credo sia sbagliato affermare che questo nuovo clima è stato ulteriormente sostenuto dal decreto sulle liberalizzazioni, che, al di là delle turbolenze che ha suscitato in alcuni settori timorosi di perdere antiche rendite di posizione, ha avuto una grande accoglienza positiva positiva nell'opinione pubblica e da parte dei principali osservatori economici, sia per la sua portata immediata, non eccezionale ma comunque significativa, sia, soprattutto, per il segnale che ha lanciato, perché si è percepito che questo Governo fa sul serio nel voler sbloccare quelle «incrostazioni» - per citare il presidente Prodi - che per troppo tempo hanno tenuto bloccato il nostro Paese. Tutti ci chiedono di andare avanti su questa strada e non può certo essere una critica accettabile quella di dire che si è fatto troppo poco. È facile rispondere che poco è comunque meglio del niente che è stato fatto in passato in tema di liberalizzazioni e che qualunque percorso inizia con un passo, purché nella direzione giusta. Credo anche che sia importante sottolineare come, già da questo provvedimento e ancor più nel DPEF, si inizi un serio percorso per ripristinare quell'equità e giustizia sociale basate su una tassazione equilibrata, ripristinando il concetto che le tasse non sono un furto dello Stato nei confronti dei cittadini, ma la base necessaria, in un Paese civile, per politiche di sostegno alla crescita, alle infrastrutture, alle politiche sociali e per una giusta ridistribuzione delle risorse secondo il dettato costituzionale. Non credo sia accettabile proseguire con un'evasione fiscale come quella che si è venuta a creare in Italia, di gran lunga la più elevata tra tutti i paesi dell'Unione Europea. Misure di contenimento dell'evasione sono la condizione necessaria, e speriamo anche sufficiente, per pensare ad una seria e duratura riduzione della pressione fiscale nel futuro. Risanamento, crescita ed equità devono e possono coesistere e crescere insieme. Il DPEF giustamente fa di queste il suo asse portante. Certo ci saranno, come è sempre stato, altri momenti per concretizzare questo progetto e in particolare, mi riferisco, alla legge finanziaria di quest'anno. L'importante è che finalmente si mette mano, come richiesto dall'Europa, ma anche da Bankitalia - tanto per citare due autorità tra le più significative - ad interventi strutturali sulla spesa pubblica, non nell'ottica dei tagli, ma in quella della stabilizzazione e del rapporto virtuoso tra crescita della spesa e crescita del PIL: pubblico impiego, pensioni, spesa sanitaria e spesa per gli enti decentrati, attraverso un nuovo patto di stabilità interna, in cui tutti si devono sentire coinvolti e resi responsabili della situazione nazionale e in cui si passi finalmente dalla logica dei tetti a quella più equa dei saldi di bilancio. Da ultimo, mi permetto di dire che sono d'accordo con coloro che sostengono l'utilità del Documento di programmazione economica, come ha fatto del resto il governatore Draghi; esso permette infatti una discussione politica ad ampio raggio, prima dei provvedimenti specifici realizzativi. Nel caso particolare, ha anche permesso, in questo inizio di legislatura, a tutti quanti, compresi coloro che come me si accostano per la prima volta da parlamentari a questo percorso politico, di comprendere nel profondo uno dei cardini fondamentali della politica nazionale: proprio il concetto di programmazione nel settore economico-finanziario, che finalmente lascia la via dell'improvvisazione e le *una* *tantum* per avviarsi all'ordinarietà, quell'ordinarietà che va intesa come virtù di chi vuole bene amministrare a vantaggio di tutti.

a votare la fiducia su qualsiasi provvedimento (avete votato più questioni di fiducia voi in questo periodo che il Governo Berlusconi, che accusavate di porre ogni volta la fiducia), ma soprattutto perché questo è un Documento di programmazione economico-finanziaria che non è condiviso, vice ministro Visco, da parte della vostra maggioranza. Non mi riferisco solo alle dichiarazioni del ministro Ferrero che non ha votato in Consiglio dei ministri questo Documento; non mi riferisco solo agli interventi che abbiamo sentito anche poco fa dei colleghi di Rifondazione Comunista, hanno detto che è un altro DPEF quello che vogliono; ma mi riferisco anche a quello che ha detto un'autorevole esponente di Rifondazione Comunista nella mia Commissione, la quale ha dichiarato di votare a favore, precisando, tuttavia, che si trattava di un voto tecnico in quanto gli obiettivi prefissati dal Governo non risultano del tutto coincidenti con l'impostazione privilegiata dalla sua parte politica, in ordine agli obiettivi di equità sociale, di tutela dei lavoratori e in generale di modello di sviluppo. Ciò significa, ministro Visco e colleghi della maggioranza, che questo è un Documento di programmazione economico-finanziaria destinato a cambiare.

che lo stesso ministro Ferrero ha auspicato la discesa in piazza dei lavoratori e delle categorie sociali, nel momento in cui non vengano rispettati o non vengano decisi all'interno della finanziaria alcune scelte che Rifondazione Comunista privilegia. È singolare vedere un Ministro che invita a scendere in piazza contro il Governo di cui fa parte, ma abbiamo assistito anche a questo.

che da quando siete andati al Governo continuate a impostare la vostra politica economica - compreso il decreto Bersani - sul fatto che avete ereditato dal Governo Berlusconi una situazione economica fallimentare.

ripresa della produzione industriale. Con tanti saluti al «declinismo» continuo di cui avete parlato durante la campagna elettorale, e dopo, solo per tentare di mascherare

Nonostante questo, non siete in grado di programmare perché si tratta di un Documento basato sulla sabbia che vi costringe a governare giorno per giorno.

Parlate sostanzialmente di rimettere in moto la concorrenza, ridimensionando in prospettiva la limitazione rappresentata dai vincoli che ostacolano la concorrenza.

dell'aumento del prezzo del carburante nel nostro Paese non è una politica sbagliata delle aziende petrolifere, ma è il sistema di distribuzione. Ciò significa che la prossima volta non saranno colpiti i tassisti, ma i benzinai, i quali già guadagnano poco, liberalizzando le pompe di di benzina e dicendo che il carburante costerà meno nel momento in cui sarà vendita non soltanto presso le pompe di benzina, ma - guarda caso - nei supermercati. supermercati. Le Coop, oltre a diventare farmacisti, diventeranno più avanti probabilmente anche dei benzinai. Tutto questo per una diminuzione della concorrenza che non porta assolutamente a niente. Ma perché, vice ministro Visco, non provate a portare la concorrenza davvero, ad esempio, nel settore del trasporto pubblico locale, che invece continua a rimanere saldamente in mano a municipalizzate che fanno acqua da tutte le parti? Come mai non provate nemmeno a liberalizzare settori di questo genere? Perché, per esempio, non impedite a certe aziende municipalizzate, nate in una certa maniera, di andare sul mercato e fare concorrenza al privato, quando sono nate per rispondere ad altre situazioni? Tutto questo non accade.

proprio ieri in quest'Aula, riducete di parecchie decine di milioni di euro la ricerca nel nostro Paese. Questo vi sembra il modo di potenziare la ricerca? Inoltre, in questo Documento ho trovato tutto sul tema

Ma davvero pensate che la maggiore attività produttiva del nostro Paese possa essere affidata al Ministero dei beni culturali? Davvero pensate che il turismo sia legato solo ed esclusivamente ad aspetti archeologici, culturali e paesaggistici? Sinceramente, credo che questa non sia la strada che porti allo sviluppo del nostro Paese:

con il quale il popolo italiano ha respinto la proposta di modifica della Costituzione che prevedeva, tra l'altro, processi di devoluzione e ritoccava in maniera significativa la già precedente modifica del Titolo V. Ciò significa Ciò significa che, ancora una volta, essendo stata archiviata - io dico fortunatamente - quella proposta di modifica costituzionale, dovrà essere affrontato il tema del rapporto fra Stato centrale e sistema delle autonomie regionali e degli enti locali. Si tratta di un problema di risorse, non solo di un problema di poteri, perché questi due aspetti sono inscindibilmente collegati tra di loro: risorse da reperire risorse da trasferire, nell'ambito di un circuito virtuoso che va ricostruito, dopo anni, soprattutto gli ultimi, nei quali molte illusioni sono state sparse a piene mani nei confronti delle autonomie, prefigurando un'immagine federale che forse, per come è stata proposta (e del resto gli italiani l'hanno respinta) nella sostanza della riforma costituzionale, non reggeva e non regge. Parlare dell'economia dei prossimi anni e del sistema virtuoso di rientro da una crisi economica profonda, che è una crisi della spesa pubblica, vuol dire anche affrontare la questione del federalismo fiscale, nonché quella di un nuovo rapporto fra Stato centrale e sistema delle autonomie. Il Documento presentato dal Governo affronta la questione del federalismo fiscale, però l'esigenza di un quadro di contenimento che certo non farà saltare dalla gioia coloro che operano negli enti locali e nelle stesse Regioni. È necessaria sempre di più, da questo punto di vista, una regia nazionale, perché lo Stato deve dare, naturalmente, il buon esempio e deve contribuire e collaborare con le Regioni e gli enti locali, affinché quei settori di recupero della spesa pubblica che vengono indicati nel Documento (la sanità, l'impiego pubblico, il sistema, appunto, delle autonomie) possano concorrere al quadro generale di risanamento non avvertendo un peso esagerato di responsabilità, ma una parte di responsabilità di un quadro più complessivo.

impegno di concertazione non burocratica, bensì di raccordo stretto con gli enti locali: qualche momento di frizione in parte già vi è stato in queste settimane ma, trattandosi

il rapporto con esse e il loro ruolo sono fondamentali per la costruzione di uno Stato diverso, capace di essere virtuoso molto più di quanto non sia stato negli anni che abbiamo alle spalle. Gli amministratori regionali e locali non vanno illusi con promesse più o meno mirabolanti, devono invece essere associati con piena responsabilizzazione, ma anche con l'invito a comprendere che operiamo in un quadro unitario verso l'Europa e non in un quadro di disgregazione

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, a primo acchito non si può dire di non condividere il quadro analitico esposto nel DPEF e gli obiettivi che vengono indicati: risanamento, crescita, equità. c'èun punto di divergenza politica ed è dato dalla configurazione di una strategia di sopravvivenza da considerare minimale. Il risanamento è affidato alla crescita del PIL, almeno per gli anni 2006 e 2007, così come prevista e in parte attuata dal precedente Governo. Entro questi margini si persegue l'obiettivo del risanamento con una procedura da «andamento lento», che volutamente ignora il punto centrale della perdita di competitività del sistema Italia e delle variabili esogene, che potrebbero aggravarne la portata e l'incidenza; una per tutte, il costo del petrolio. Dopo aver condotto una campagna elettorale che dalla denuncia catastrofica del Governo allora in carica faceva derivare l'annuncio quasi miracoloso della ripresa e del rilancio («la macchina riparte» era lo *slogan*), assistiamo a una prospettazione, che ho già definito minimalista. La macchina continua ad andare così come stava andando. Il Governo Prodi si attiene alla linea molte volte sperimentata dello stellone,

resisteva a tutti i tentativi e alle richieste di programmazione del centro-sinistra, affidandosi soltanto a una doppia scelta: il Governo della congiuntura e lo stellone, che avrebbe consentito la ripresa. Eppure sono stati anni in cui l'Italia è cresciuta quasi dell'8 per cento, ma questo argomento serve soltanto per gli storici. Il DPEF non può però non evidenziare che la ripresa è affidata esclusivamente alla tenuta ed all'incremento della domanda interna. Quanto alle esportazioni è ovvia la constatazione che la perdita di competitività in uno alla perdita costante di produttività - perché questo è il nesso che sfugge totalmente al DPEF - non assicura la prospettiva, largamente sperimentata in passato, che un rilancio delle esportazioni divenga il motore principale dello sviluppo; allora bastava un'intensificazione, un'accelerazione del moto della locomotiva tedesca per godere di un traino. Non sarà corrispondente al vero la tesi del declino, però oggettivamente assistiamo a un ridimensionamento del sistema produttivo italiano, addirittura ad un'uscita da settori importanti e decisivi rispetto al futuro e soprattutto continuiamo a sopportare il il peso dell'impotenza nel settore energetico. Il DPEF traccia un profilo minimalistico sul piano degli obiettivi concreti della crescita; è assolutamente privo dell'indicazione e precisazione degli strumenti. Sulle linee del risanamento, rimanendo all'interno della logica dell'esistente, è ovvio che, come preme sottolineare allo stesso ministro Padoa-Schioppa, sui saldi e sulle cifre non ci sia disaccordo di fondo, tuttavia l'UDC, e penso l'intero schieramento di opposizione, lo dico al Ministro del tesoro per la dichiarazione di questa mattina, non potrà essere d'accordo con la legge finanziaria in quanto coerente proiezione del DPEF. Sulla politica finanziaria ed economica la maggioranza che esprime l'attuale Governo aveva annunciato una discontinuità, anzi questa parola continua a riecheggiare ripetutamente in questa Aula. Di fatto, però, Padoa-Schioppa e Prodi stanno sul sentiero di Tremonti, che pure aveva uno scenario dell'economia internazionale diverso, ma ne riducono la larghezza. Infatti, ed è paradossale, la preoccupazione predominante di questo DPEF, e forse non potrebbe non essere diversamente, è il risanamento, soltanto in via successiva la crescita, e anche qui non si vede la discontinuità promessa. Il risanamento però, onorevoli senatori, ha un vincolo assoluto. Il debito è collocato sul mercato internazionale per una grande parte, credo quasi il 60 Il relativo costo, che è stato una leva assai importante nella possibilità di riduzione in altri tempi anche al momento dell'addio dell'euro, oggi è rigido. E qui si assiste alla esercitazione pirotecnica anche di questi giorni. Si additano come obiettivo da colpire alcune posizioni di rendita e non si possono indicare le rendite finanziarie. Tutta la polemica ideologica, e non anche di dottrina, contro le rendite trova il ripiego sui tassisti e sui ceti medi. Mi pare che Ricolfi sulle colonne de «La Stampa» abbia bene precisato cosa si debba intendere per rendite in Italia e abbia dimostrato che le rendite attraversano tutti i ceti sociali. Ricardo e Marx servono allora a poco a leggere questa realtà. Il risanamento che si ipotizza ha una incognita molto conosciuta - mi si perdoni l'ossimoro - la spesa pubblica e qui il Governo è atteso alle scelte che con la legge finanziaria proporrà in ordine a pensioni e sanità; saranno problemi seri per la maggioranza? Non credo che l'alleanza con i borghesi buoni potrà avere tenuta e un qualche avvenire. Questo DPEF allora nella scrittura gentile di una trama più complessa, è il manto steso sulle contraddizioni di questa maggioranza e soprattutto sulle reticenze e sui silenzi. Ho detto delle incognite sulla sanità e sulla previdenza, ma mi chiedo, qualcosa sulle strategie per il controllo e la ristrutturazione della spesa in ordine all'intero sistema della pubblica amministrazione, e cioè il controllo della spesa degli enti locali periferici? Non credo che la maggioranza di centro‑-inistra sia in condizione di intaccare il sistema consolidato di alcune Regioni, soprattutto quelle del Centro-Italia. È poi scarsamente credibile tutta la proiezione della pressione fiscale perché da un lato si enfatizzano le misure per l'equità e quelle miranti al recupero dell'elusione e a prevenire comportamenti fraudolenti, dall'altra si indica una stabilizzazione della pressione fiscale sostanzialmente attorno al 41 per cento, nonostante i conclamati recuperi di basi imponibili senza verificare una adeguata redistribuzione di risorse disponibili. Sulle politiche fiscali il centro-sinistra preferisce il mezzo dell'oppressione fiscale piuttosto che quella della leale collaborazione tra Fisco e contribuenti e sulla via della giustizia fiscale non si dice alcunché in ordine ad una impostazione che, proprio per iniziativa dell'UDC, si fece largo nella passata legislatura e viene riproposta in questa che riguarda la riforma della tassazione della famiglia con l'introduzione del quoziente familiare. Qualche osservazione poi devo fare nel merito delle strategie di attuazione di una politica economica di sviluppo. Sulle privatizzazioni credo che il Governo non abbia più il tesoro di famiglia che è stato già abbondantemente Sulle liberalizzazioni, dopo il can can di questi giorni, quando il Governo presenterà qualcosa di efficace per attuare politiche di concorrenza effettiva e concreta, per esempio, sulle tariffe elettriche e sulle tariffe telefoniche? Sulla ricerca, quando strumenti concreti per coordinare, intensificare e sviluppare un'area che è decisamente carente nel nostro Paese? Sugli investimenti produttivi, mi limito ad una sola osservazione. Nel DPEF è indicato un accenno al settore agroalimentare. Ma il Governo è consapevole dei problemi attuali? È saltato il negoziato dell'UTO, ma l'Unione sta procedendo ad una proposta delle singole organizzazioni di mercato a partire, per esempio, da quella del settore vitivinicolo in termini malthusiani, con la proposta di riduzione di 400.000 ettari del vigneto in Europa. Sulle infrastrutture, la mancanza di ogni decisione sulle posizioni interne alla maggioranza in ordine alla TAV, al corridoio 5, al MOSE, al ponte di Messina, ha indotto - ho ascoltato poc'anzi l'intervento del senatore Brutti - ad un forte richiamo. Ovviamente non condivido la proposta del senatore Brutti di utilizzare le risorse per ora appostate per il ponte sullo Stretto per la copertura finanziaria di questo elenco di opere. Circa il Mezzogiorno, esso ormai è rimesso esclusivamente alle poche righe del paragrafo V «Strategia per la competitività e il riequilibrio territoriale» e quindi esclusivamente agli spazi da definire all'interno del quadro strategico nazionale. Se l'Unione Europea dà un po' di soldi, questi valgono per il Sud. Quanto è lontana la legge n. Tutti i proclami sulla centralità della questione meridionale sono finiti in un cassetto del dimenticatoio. Certamente vi è una questione settentrionale e va anche bene l'incontro di Milano di ieri, purché questo non risponda innanzitutto a tattiche politico-elettorali minori. Ma il problema del Sud, dalla coalizione del centro-sinistra, che proprio al Sud ha vinto le elezioni, credo non possa essere gettato alle ortiche. Mi chiedo, poi, quanto incidano sul piano della politica le rappresentanze del Sud stesso, stando a quello che leggo nel DPEF. Vedo, poi - e riprendo l'argomento - archiviata la questione o meglio il progetto del ponte, che invece non deve essere archiviato. Anche per questi ultimi e specifici motivi, da parte di un'opposizione come quella dell'UDC non può venire consenso al DPEF.

sta ascoltando tutti gli interventi in un'Aula piuttosto deserta. Dico subito che condivido l'impostazione generale del Documento e che il mio voto sarà favorevole. Questo, però, non mi impedisce di interloquire con il Documento di programmazione economico-finanziaria considerandolo anche come occasione privilegiata, nella quale il Parlamento offre al Governo indicazioni e orientamenti per la finanziaria. In quest'ottica, avanzo una prima osservazione. Sarebbe stato preferibile attendere qualche altro giorno per poter affrontare e per poter offrire un quadro progettuale più preciso. Mi riferisco al quadro strategico nazionale 2007-2013, di cui si dice espressamente nel Documento che sarà definito entro l'estate. Mi riferisco anche all'allegato delle infrastrutture, che oggettivamente non contiene le scelte e le priorità che gli stessi ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, Di Pietro e Bianchi, si sono impegnati a presentare al Parlamento subito dopo l'estate. Ciò oggettivamente non ci consente di affrontare in modo approfondito la questione del Mezzogiorno. intendo trattare questo aspetto, che è oggetto di particolare attenzione nella risoluzione con cui la maggioranza approverà il DPEF, come espressione di interessi territoriali, ma come questione che attiene all'interno Paese, nella convinzione che il Sud rappresenti una priorità e un'opportunità per l'Italia intera e per il suo sviluppo. Condivido, dunque, gli obiettivi che il DPEF individua, nella consapevolezza che essi sono organici ad una politica di sviluppo del Mezzogiorno, di cui, però, è opportuno precisare alcune modalità che meglio ci consentano di perseguire gli stessi. Occorre innanzitutto riprendere in considerazione il tema della fiscalità di compensazione. In tal senso, chiedo espressamente al Governo di riaprire un confronto con la Commissione europea, anche alla luce dell'articolo 87, comma 3, lettera *a)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, che con chiarezza recita: «Possono considerarsi compatibili con il mercato comune: agli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione»; e, ancora, alla lettera *c)*: «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse». in considerazione anche il Regolamento che la Commissione ha approvato per quanto riguarda i fondi strutturali dal 2007 al 2013, si dice con chiarezza

a condizione che questi aiuti siano limitati nel tempo e decrescenti. Il Parlamento europeo, in una risoluzione del 14 febbraio 2006 - che anch'io ebbi di votare - ha dichiarato espressamente «l'introduzione di condizioni fiscali vantaggiose per periodi transitori non superiori a 5 anni » può essere«funzionale ad un approccio più efficiente alla concessione di aiuti regionali». Dunque, vi sono strumenti che ci consentono di riprendere con forza questa prospettiva. A coprire l'onere di un fiscalità compensativa potrebbero contribuire anche il risanamento del lavoro irregolare e sommerso e un buon recupero dell'evasione fiscale. Queste somme potrebbero essere prioritariamente destinate proprio alle zone dalle quali sono state recuperate. Del resto, occorre convenire che la minore presenza ed efficienza di servizi pubblici in alcune Regioni meno sviluppate produce oggettivamente disuguaglianze anche economiche tra le imprese e che, perciò, una fiscalità differenziata non violerebbe affatto i principi della concorrenza. Altro punto fondamentale è quello relativo a un nuovo sistema di trasporti e infrastrutture nel Mezzogiorno. È un punto nodale di quanto il programma dell'Unione prevede per il Sud. L'allegato delle infrastrutture sostanzialmente fotografa la situazione esistente ma, prima che il piano per la mobilità interna e per le infrastrutture sia presentato,

È necessario invece operare delle scelte macro e interregionali che facciano sistema e che siano organiche ad uno sviluppo reale del Sud e dell'intero Paese, Paese, coinvolgendo le Regioni, che non beneficiano soltanto se l'opera è realizzata sul proprio territorio. Del resto, non si può più tollerare che per i trasporti al Sud siano utilizzati esclusivamente o quasi fondi europei, mentre diminuisce la spesa ordinaria. Occorre invece concentrare più fondi statali per le infrastrutture al Sud e impiegare in larga parte risorse private per il Nord. La già richiamata necessità di definire strategie condivise rende accettabile la proposta giunta dai presidenti delle Regioni del Sud, dai sindacati confederali e da Confindustria di istituire un organismo leggero, una sorta di agenzia tecnica, per lo sviluppo dei trasporti e della logistica nel Mezzogiorno, in cui sia rappresentato lo Stato, le Regioni, le Ferrovie dello Stato e l'ANAS, con il compito di coordinare gli investimenti e assicurare un sistema di pianificazione e controllo. Attenzione particolare va data inoltre ai sistemi urbani del Sud, un Sud nel quale spesso le regole del governo del territorio sono state dettate esclusivamente dalle emergenze di varia natura, da quelle ambientali, a quelle idrogeologiche, a quelle economiche e sociali. Occorre invece considerare i sistemi urbani come uno snodo centrale nelle politiche di coesione e di competitività per gli obiettivi di Lisbona. Occorre passare dal degrado allo sviluppo; lo stesso regolamento comunitario sul Fondo sociale europeo, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sul Fondo di coesione individua questa come priorità assoluta nella pianificazione dello sviluppo regionale. Ciò renderà certamente più agevole orientare da parte del Governo un'azione particolare verso una questione centrale per il Sud. L'esperienza dei contratti di quartiere avviati nel 1998 è stata nel complesso positiva, ma il ritardo è sotto gli occhi di tutti. Lo stesso programma Urbano, pur avendo interessato dal 1994 al 2006, città del Mezzogiorno è rimasto un programma fondato su progetti pilota che fungono più da modelli virtuosi che da reali elementi di trasformazione del territorio. Non mancano altri strumenti finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come il programma Sistema che interessa otto aree territoriali del Sud,

le risorse in modo efficace su un progetto organico per le aree urbane del Sud. L'ultima riflessione è che il cuneo fiscale deve seguire in qualche modo una distinzione territoriale. In ultimo, dico ai colleghi che parlare del Sud in modo specifico non significa avere un'idea settoriale degli interventi; parlare del Sud e impegnarsi per esso significa impegnarsi per l'intero sistema Italia,

Signor Presidente, colleghi e colleghe, rappresentanti del Governo, signor Ministro, innanzitutto vorrei esprimere il mio positivo giudizio sull'impianto generale del DPEF, ed in particolare sull'esigenza di coniugare strettamente risanamento e sviluppo con l'equità sociale. Così come è condivisibile l'obiettivo di diminuire il tasso di disoccupazione ed aumentare quello dell'occupazione in particolare dei giovani, delle donne e dei cosìdetti lavoratori anziani. anziani. Sono d'accordo che per il nostro Paese sia indispensabile affrontare contemporaneamente il problema della perdita di produttività e competitività così come quello della garanzia della piena occupazione. Va però precisato da questa maggioranza e dal nostro Governo che la perdita di competitività del nostro sistema, che investe sia il settore della produzione manifatturiera sia quello dei servizi, non è assolutamente imputabile ai lavoratori che in questi anni invece hanno visto progressivamente peggiorare le loro condizioni economiche e sociali, i loro diritti; mentre è costantemente aumentata la produttività delle prestazioni lavorative. lavorative. Ritengo debba essere affermato con estrema chiarezza che non esiste nel nostro Paese alcun problema di costo del lavoro. Anzi, va evidenziato, come ci dicono le statistiche, che il costo del lavoro in Italia si colloca agli ultimi posti nella graduatoria (siamo al dodicesimo!) e nelle ultime posizioni, se ci si rapporta con i Paese maggiormente industrializzati a livello mondiale. Per questo, ho difficoltà a comprendere e condividere pienamente la proposta di riduzione di cinque punti del cuneo fiscale per la parte relativa alle aziende. Si continua così di fatto ad operare scelte di politica economica già vissute, sulla scia di quelle compiute negli ultimi decenni, nel senso di continuare a ridurre il costo del lavoro per le imprese che non hanno prodotto né sviluppo né competitività, ma anzi hanno contributo fattivamente all'attuale rovinosa situazione economica del nostro Paese. Nondimeno, mi preme evidenziare positivamente la discontinuità che nel DPEF si manifesta su questa materia, in primo luogo perché esclude interventi di taglio sugli oneri previdenziali, in secondo luogo perché l'orientamento è quello della selettività nei confronti delle imprese, in particolare nei confronti delle imprese che assumono lavoratori a tempo indeterminato. Nel Documento si afferma il principio che una parte della riduzione dovrà avere come beneficiari i lavoratori, senza però alcuna specificazione; a questo proposito, ritengo necessario che vada operata una scelta che, per quanto mi riguarda, veda il beneficio per i lavoratori non inferiore al 50 per cento della riduzione del cuneo, in modo tale da garantire un aumento salariale immediato. Signor Presidente, esiste ormai nel nostro Paese una questione grande come una casa che si chiama «questione salariale», ed infatti nel corso degli ultimi tredici anni è stata operata un'enorme rapina, a tutto vantaggio della rendita finanziaria e del grande capitale, e ad esclusivo danno dei redditi da lavoro che hanno registrato una costante perdita, aggravata anche dalla progressiva riduzione delle tutele sociali, delle prestazioni assistenziali e previdenziali; dalla vertiginosa impennata dei prezzi al consumo, delle tariffe, delle spese per l'istruzione, per le cure sanitarie, per la casa ed i trasporti. È tornata, dopo decenni dalla sua scomparsa, la cosiddetta sindrome della quarta settimana, in virtù della quale, pur lavorando, il salario non è più sufficiente. Secondo i dati forniti da Bankitalia, sono circa sei milioni e mezzo i lavoratori che guadagnano meno di mille euro al mese e circa 10 milioni di pensionati che ne guadagnano meno di 800! Gli ultimi dati confermano che dal 2002 al 2005 il lavoratore dipendente tipo ha cumulato una perdita di 1.647 euro, di cui 1.082 imputabili alla cosiddetta politica della concertazione o dei redditi, come la si voglia chiamare, e di altri 575 imputabili alla mancata restituzione del *fiscal drag*. Occorre invertire la rotta, affrontando il tema della redistribuzione della ricchezza prodotta dal Paese, sottraendola alla rendita finanziaria per restituirne una quota consistente ai lavoratori dipendenti, gli unici, a mio parere, che producono ricchezza. Per questo è indispensabile la reintroduzione di un meccanismo automatico di rivalutazione delle retribuzioni e dei salari, sicuro elemento di giustizia sociale e di difesa dei settori più deboli. Ripristinare la scala mobile vuol dire tornare ad avere salari in grado di reggere i colpi del carovita, uscendo dall'assurda situazione che vivono oggi i lavoratori, costretti a scioperare per ottenere una parziale restituzione di quanto perso a causa dell'inflazione. Ne deriverebbe, conseguentemente, anche una rivalutazione del ruolo e delle funzioni sia del contratto nazionale sia della contrattazione di secondo livello. Altro capitolo assai delicato del DPEF è quello concernente le pensioni; infatti, se da una parte si deve apprezzare l'intendimento di ridurre il famigerato scalone del 2008, dall'altra non si può non essere preoccupati per alcune indicazioni contenute che individuano nella revisione dei limiti di età o dei coefficienti di trasformazione possibile terreno d'intervento. Per quanto mi riguarda, queste scelte sono assolutamente non condivisibili anzi, inaccettabili e quindi, se recepite nella prossima finanziaria, troveranno la mia più ferma contrarietà, con i conseguenti comportamenti. Sull'aumento dell'età pensionabile, l'unica via valida come soluzione percorribile è quella della volontarietà, eventualmente incentivata, per altro già prevista dalla C'è poi un problema vero da affrontare, e possibilmente da risolvere, che è quello relativo all'imponente perdita di potere di acquisto dei redditi da pensione, in particolare per quelli più bassi. S'impone dunque in tempi brevi, così come è previsto nel programma, l'identificazione di un nuovo meccanismo di indicizzazione delle pensioni al costo della vita, la restituzione del *fiscal drag*, tutto ciò unitamente ad altre iniziative di equità fiscale che permettono di garantire ai pensionati, così com'è previsto dalla Costituzione, una vecchiaia dignitosa. Non è solo una questione di giustizia sociale, bensì anche una precisa scelta di politica economica anticiclica. Se oggi infatti - vivaddio - nelle tasche delle famiglie italiane entrassero 200 euro in più al mese, certo non si risolverebbe il problema del declino, ma probabilmente si risolverebbe quello della stagnazione della domanda. Nel programma dell'Unione si afferma poi la volontà di superare la precarietà e la legge n. Personalmente continuo ad essere convinto che questa non sia una legge riformabile e che debba essere abrogata nella sua totalità. Ciononostante, un intervento minimo necessario ed urgente potrebbe indicarsi nell'affiancare al superamento dello *staff leasing* e del lavoro a chiamata - le uniche due tipologie di lavoro individuate l'impegno a rivedere radicalmente e da subito la normativa dei rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale nonché quelle sui portatori di *handicap* e sui soggetti svantaggiati. È apprezzabile poi la decisione di aumentare i contributi previdenziali per i cosiddetti lavoratori atipici a carico delle imprese.

questo delicato tema ritengo che si sarebbe potuto e dovuto osare di più. Il nostro programma si pone l'obiettivo di rendere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato la norma, sull'indispensabile presupposto che il lavoro flessibile e precario costi quantomeno come quello a tempo indeterminato ed il lavoro atipico e flessibile possa usufruire dei medesimi diritti e delle medesime tutele. Fino a quando questi fondamentali obiettivi non saranno raggiunti, e quindi i relativi principi compiutamente affermati, la triste condizione dei precari a vita di vedersi negata la possibilità di costruirsi un futuro continuerà inesorabilmente inesorabilmente ad aumentare. Sempre a questo proposito, e sempre con l'intenzione di ridare valore e dignità al lavoro e mezzi sufficienti ai lavoratori per condurre una vita dignitosa, e di mettere la pubblica amministrazione nelle condizioni di erogare servizi di qualità nel pieno rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, oltre agli interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse già previsti, sarebbe opportuno un provvedimento governativo di carattere generale volto a ridurre e superare le forme di precariato nell'ambito della pubblica amministrazione. Infatti, negli ultimi due anni le misure di blocco del *turn over* nel

indeterminato, ma anche perché tale intervento non comporterebbe alcun costo aggiuntivo per le amministrazioni interessate.

è la prima volta che prendo la parola in quest'Aula. Quindi, un saluto caro e cordiale a tutti e a ciascuno, a partire da lei, signor Presidente.

in cui vengono concluse le discussioni, consenta veramente al parlamentare

sarà nuovamente praticata da qui a qualche giorno. Mi chiedo, al di là del problema, signor Presidente, Presidente, della compatibilità con la norma costituzionale, se non erro con l'articolo 94 della Costituzione, se questo non si traduca in una detrazione, in una sottrazione delle prerogative del parlamentare. Mi pare che il tutto possa tradursi così, signor Presidente: bene, dedichiamo uno spazio di tempo alle osservazioni; ognuno è libero di avanzare ed esprimere le proprie opinioni, dopodiché, sul Documento, su cui tutti hanno avuto possibilità di interloquire e di dire, il Governo pone la fiducia. A

cercare di stabilire un dialogo, un incontro, un confronto nell'Aula parlamentare se tanto la sorte di tutto ciò che avviene ha un esito scontato? La fiducia sul proprio Documento! Credo, signor Presidente, che nessuno in Aula

che definisce come "doppia frenesia" quel moto per cui, dopo essere andati freneticamente in un senso, si va o si deve andare freneticamente in senso opposto. Questo varrebbe per l'attuale maggioranza e per l'attuale minoranza. Non credo però che in entrambi ci sia questa doppia frenesia. Allora, diamoci una regolata, signor Presidente! Rendiamo possibile la partecipazione di tutti e di ciascuno alle elaborazioni parlamentari. A questo punto, A questo punto, potrebbe avere fondamento il sospetto che ieri il senatore Andreotti con linguaggio consono al suo rilievo personale e storico

Credo che il senatore Andreotti, con tutta la riservatezza e la prudenza del linguaggio che è tipica dell'uomo, volesse andare oltre, signor Presidente, e intendesse dire che, soprattutto in regime bipolare, non è possibile, sulla base di una consuetudine, prescindere dal fatto che la nostra Carta costituzionale prevede la fiducia una e una sola volta per il Governo, e che la stessa norma la sfiducia su mozione, ma non una fiducia ripetuta e tematica! A questo punto, dal il senatore Andreotti ha voluto essere un po' ermetico, io, che non ho la sua virtù, vado oltre e dico: signor Presidente, è un problema, quello della liceità e della costituzionalità del ricorso alla fiducia, che dovete porvi. Ve lo dovete porre alla luce della norma, non alla luce della giurisprudenza di fatto, di fatto, creatasi sulla base di una cattiva applicazione della norma costituzionale per mezzo secolo.

limitarsi agli inviti, alle sollecitazioni di prudente atteggiamento e di buon dialogo.

una regolata; non è possibile un'Aula parlamentare dove la regola è lo scontro del muro contro muro. Vorrei approfittare di una considerazione recentissima, di qualche giorno fa, del solito, puntuale Padre Simone de "La Civiltà cattolica", che definisce l'attuale momento nel modo seguente. Dice «La Civiltà Cattolica», signor Presidente, che, nonostante le attuali difficoltà nei rapporti tra maggioranza e opposizione, e tenendo presente che in autunno i lavori parlamentari saranno assorbiti quasi completamente dalla discussione della legge finanziaria, è auspicabile che il ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, Vannino Chiti, forse insieme ai Presidenti delle Commissioni parlamentari affari costituzionali, ricerchi costituzionali, ricerchi le necessarie convergenze innanzitutto sul metodo da seguire, per un dialogo effettivo e costruttivo fra maggioranza e opposizione, partendo dal tema della riforma costituzionale. Il problema, caro Presidente, sul tappeto è quello della riforma costituzionale. Chi le parla

Lo avvertono anche quelli de "La Civiltà Cattolica" che, certo, non sono vicini alla mia parte, né al centro-destra; semmai, da Bartolomeo Sorge a Padre Michele Pisani e ad altri, sono piuttosto vicini alle vostre posizioni culturali e politiche. Allora, Presidente,

È un vostro diritto tentare di costruire consenso elettorale a Milano, però tenete conto che Milano è una città che ha fortemente radicati i suoi principi, le sue aspettative, la sua volontà di città laboriosa, autonoma, libera e democratica. Non si lascerà incantare dalle continue missioni di pace; occorre che si sia effettivamente costruttivi nei rapporti. Incominciamo da quest'Aula. Chi fa ostacolo

oggi pensa di non potersi moderare, chi crede, al vostro interno, di poter andare avanti a colpi di fiducia,

la governabilità di questo Paese, vi diciamo che il nostro ruolo parlamentare è in funzione delle aspettative del Paese. Quanto al DPEF, signor Presidente,

Io mi chiedo, ma se lo sono chiesti tutti quelli che si sono occupati del DPEF, come sia possibile parlare di sviluppo di equità se le condizioni da voi previste di crescita sono così minimali e, peraltro, regressive per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011. Mi chiedo come sia possibile che non si tenga conto del fatto che questa crescita ponderata di PIL è prevista soltanto attraverso la domanda interna, e non vi sia nessun concorso, in termini di crescita, della domanda esterna e internazionale.

Fra le tante cose, afferma in modo quasi sibillino che: «Il Governo intende proseguire la liberalizzazione dei servizi energetici.» - ci mancherebbe altro che fosse diversamente

per fruire della *golden share* dello statuto dell'ENI, per cui noi perderemmo automaticamente e conseguentemente L'ENI. a concludere, senatore Fruscio. al fatto che lei ha utilizzato i tempi residui del Gruppo della Lega Nord, mentre in un primo momento era stato detto che il suo intervento avrebbe avuto una durata di dieci minuti.

il relatore di minoranza, senatore Baldassarri, questa mattina ha accusato la sinistra radicale di acquiescenza alle politiche dell'Ulivo e per derivazione diretta, con un sillogismo le cui premesse andrebbero verificate, alla grande finanza. Personalmente, non ricordo che il Governo Berlusconi, di cui Baldassarri era ascoltato vice ministro, si sia contraddistinto come campione dei deboli contro i forti. Non ricordo nemmeno che le politiche economiche del Governo di centro-destra siano state caratterizzate da particolare fermezza nei confronti di un mondo finanziario del quale l'ex Presidente del Consiglio era ed è parte integrante, non corpo estraneo. Anzi, il Governo Berlusconi è stato impotente nei confronti di una finanza d'assalto che ha speculato ai danni di milioni di cittadini, lavoratori, risparmiatori: Parmalat, Cirio, Banca di Lodi, furbetti del quartiere, le stesse vicende Unipol e Fazio, per non parlare di scalate poco chiare come quelle del «Corriere della Sera», sono lì a testimoniare come banche, assicurazioni, società immobiliari e multinazionali quotate in borsa, negli ultimi anni, in Italia pensavano di operare in un contesto a maglie larghe, in cui i controllori e i i garanti chiudevano uno o entrambi gli occhi e la politica non tutelava i cittadini; nel quale una supponenza, che spesso si traduceva in un'autoconvinzione di intoccabilità, era indice di una tranquillità che il sistema politico, evidentemente, nel suo complesso garantiva. Questa stagione, per quanto ci riguarda, è finita: un diverso spirito pubblico va trasmesso al Paese. Non è un caso che il DPEF sia così analiticamente attento al rigore, alla legalità fiscale, al rispetto dei trattati europei e degli impegni con gli elettori, alla modernizzazione della pubblica amministrazione, alla revisione dei criteri di costruzione del bilancio. È un DPEF che non fa ricorso ad espedienti temporanei, come le *una tantum,* o rozzi e inefficaci come i tetti di spesa. C'è un'ansia da *civil servant* nel ministro Padoa-Schioppa, che noi abbiamo percepito e apprezziamo: recuperare un alto senso dello Stato e delle istituzioni non è fatto politico secondario. Esso però non è sufficiente e il dissenso all'interno del Governo va letto in questo senso generale: il risanamento del Paese non è solo un fatto tecnicoo etico. La costruzione di un bilancio non è semplicemente la soluzione di un'equazione a molte incognite, né la complessità sociale ed economica può essere ricondotta unicamente ad un quadro sinottico matematico, per quanto ben costruito. Lo stesso articolo di Luigi Spaventa, apparso oggi su «la Repubblica» e citato dall'opposizione a sostegno delle proprie posizioni si conclude con la presa d'atto che l'attuale DPEF, stabilito il saldo netto da finanziare dal bilancio dello Stato per il 2007 a 29 miliardi, va considerato nella sostanza un impegno economico di legislatura che non può e non vuole chiudere le scelte del Governo e del Parlamento in una rigida cornice numerica. Del resto, che sarebbe esercizio vano lo dice l'oscillamento dei prezzi del petrolio e delle materie prime. Le posizioni dialogiche del ministro Ferrero, quindi, hanno lasciato aperto uno spazio politico a beneficio di tutti per proseguire un confronto allargato, spazio che a nostro avviso è già stato positivamente ridisegnato dalle rappresentanze economiche, sociali e politiche. Del resto, per fare solo un esempio che però crediamo significativo, la drastica affermazione del Governatore della Banca d'Italia sulla necessità di alzare l'età pensionabile non ha riscontro nell'analisi del DPEF, nel quale si afferma che la spesa pensionistica ha registrato una dinamica relativamente più contenuta rispetto a quella di altre voci di spesa. Essa è pienamente sotto controllo e il suo incremento rispetto al livello del 2005 sarà nel 2040 di soli 1,2 punti percentuali (come si evince da pagina 126); i conti per lo Stato sono destinati a migliorare con la lotta al lavoro nero, la regolarizzazione dei lavoratori migranti e, in più lunga prospettiva, il potenziale aumento della natalità sempre grazie al contributo degli immigrati. Con intelligente oculatezza il Ministro oggi pensa di puntare sulla volontarietà dell'innalzamento dell'età pensionistica e non ad interventi legislativi. Con la risoluzione che tra poco voteremo il confronto trova una sua prima e positiva sintesi in attesa della finanziaria. L'impegno sui saldi, descritto analiticamente nel DPEF e ripreso dalla risoluzione, sarà mantenuto coniugando lavoro e impresa; giustizia sociale e crescita; ambiente e sviluppo; diritti universalistici costituzionali e risanamento; pubblico e privato.

il cuneo, gli interventi sulla spesa pubblica, le misure per il rilancio del sistema produttivo e delle politiche sociali, la valorizzazione dell'istruzione e della cultura e una lotta rigorosa alla criminalità organizzata. E queste scelte vanno lette anche con con lenti che non siano solo quelle del PIL, cioè di una crescita della ricchezza complessiva del Paese misurabile con una calcolatrice. Signor Presidente, signori del Governo, tra il luglio 2004 e il giugno 2005 due famiglie su tre in Italia si sono dichiarate soggettivamente povere (indicatori ISAE, pagina 87 del Documento di programmazione economico-finanziaria). Sarà questo il primo grafico che andremo a vedere tra cinque anni: se l'indicatore sarà in netto calo, obiettivo per cui lavoreremo con tenacia, la difficile sfida che oggi lanciamo a noi stessi, all'opposizione e al Paese, sarà stata vinta.

nel verificare come questo DPEF arriva in Aula, penso vada sottolineato anche l'ultimo intervento del collega Albonetti, il quale, nel contestare il nostro collega Baldassarri, credo abbia detto cose inesatte: ha elencato una lunga serie di scandali

il lavoro su tale provvedimento. Tornando al DPEF, mi stupisce leggere nell'introduzione - e se non si trattasse di una cosa seria farebbe anche sorridere - la premessa tecnica a questo Documento. Vi è un capitolo intero intero dedicato al contesto economico internazionale e alla relativa congiuntura economica, quella stessa congiuntura che durante il Governo Berlusconi per l'allora opposizione non esisteva e non poteva mai essere presa neppure a parziale motivo delle difficoltà di rilancio economico del Paese. Oggi invece è premessa a tale Documento; questa quindi è la prima bugia, la prima falsità di tutto quello che ci siamo sentiti dire addosso nella precedente legislatura. Siccome questo provvedimento, oltretutto,

la pretesa di indirizzare i Documenti di programmazione economica e finanziaria dei prossimi cinque anni. In esso si parla di sviluppo, risanamento, equità; ma di questi tre punti, sicuramente condivisibili,

Direi che tali filosofie, pur condivisibili, non le troviamo, facciamo proprio fatica a trovarle in tutta la politica del Governo. Un DPEF perciò che non dà affatto risposte in questa direzione. L'approccio del Documento, oltre a essere particolarmente pessimista sul quadro attuale della domanda di mercato interna e estera, contraddice ancora una volta le posizioni dell'Unione, che fino a qualche settimana fa le quali per una buona politica economica non si sarebbe in grado di incidere sugli andamenti dell'economia reale con provvedimenti come il DPEF. Questa è una rinuncia a tutto campo

Ma come, proprio nella fase storica in cui i Paesi emergenti dell'Est europeo entrano in Europa a pieno titolo e guardano al modello italiano e, in particolare, a quello del nord-est fatto di una rete diffusa di piccole e medie imprese, l'Italia da il primo colpo di scure a questo modello, prima con il decreto Bersani, ed abbandona quegli strumenti di difesa, soprattutto dalla concorrenza estera, proprio in questo DPEF? Il DPEF sconta, da questo punto di vista, le conseguenze dell'allarmismo sullo stato dei conti pubblici che ha contraddistinto l'avvio dell'attività del nuovo Governo. appena insediato e senza ancora disporre di un quadro aggiornato sulla effettiva situazione dei conti pubblici, il Presidente del Consiglio e lo stesso Ministro dell'economia si sono distinti per un eccesso di zelo nel denunciare un presunto e non dimostrato stato di grave criticità della finanza pubblica. Noi, invece, diciamo che occorre riprendere quel percorso di sostegno alle nostre imprese che preveda una visione chiara del ruolo che l'Italia può e deve svolgere sui mercati internazionali, l'Italia dell'ingegno, della creatività, della tipicità, del *made in Italy*. Attorno a queste direttive vanno ridisegnati i provvedimenti di fiscalità selettiva, di agevolazione per i trasferimenti generazionali, di sostegno a questa crescita dimensionale. Credo che fareste bene a sentire quali sono gli umori, in particolare, del Nord-Est (in cui io sono stato eletto) delle categorie di fronte a questi provvedimenti, caro Ministro. L'impressione che si trae dalla lettura del Documento è che in realtà non sia il rafforzamento dei tassi di crescita l'obiettivo che prioritariamente sta a cuore a questo Governo, quanto piuttosto solo ed esclusivamente - come ricordavo all'inizio del mio intervento - quello del risanamento, e basta. Il risanamento ci può andare bene ma non può bastare, soprattutto non può bastare all'economia del Paese. Sono evanescenti le politiche sull'incentivazione delle pari opportunità su questo Documento. Anche per quanto riguarda l'occupazione giovanile vengono spese poche righe disgiunte, addirittura, da una visuale che inserisca in una politica della famiglia il futuro dei figli. Risulta poi evidente come questo Governo sia privo di una chiara linea sugli investimenti infrastrutturali fondamentali per lo sviluppo del Paese. Il Documento si limita a osservare come sia necessario operare, attraverso una razionalizzazione, gli interventi in base ad alcune priorità, senza definire l'impegno finanziario che intende assumere.

Vediamo però che il Ministro per le infrastrutture un giorno c'è e un giorno non c'è. Nel frattempo il Presidente del Consiglio va a Milano a parlare di infrastrutture, non si capisce a titolo di quale Ministro, visto che il ministro in quella fase si era auto sospeso. E ancora, poche righe dedicate al sistema agroalimentare - lo ha ricordato anche il collega Scarpa Bonazza Buora - veramente poche che rappresentano la conferma di una scarsa attenzione nei confronti di questo comparto fondamentale nel traino dell'economia del Paese. Emerge poi con chiarezza un altro dato molto preoccupante: la totale scomparsa del tema delle privatizzazioni. Forti perplessità suscita anche la riflessione inserita nel Documento sul sistema pensionistico, posto che da una parte si afferma la necessità di allargare la base contributiva per mantenere in equilibrio il sistema e dall'altro si afferma che per abbassare lo scalone previsto dalla riforma vigente sarebbero necessarie risorse ingenti ma non si specifica da dove verranno prelevate e quante siano queste risorse. In conclusione, siamo in presenza di un Documento carente negli obiettivi e poco credibile nei numeri e nelle strategie per raggiungerli. Questa mattina, forse perché era molto presto, il Presidente della Commissione ricordava come questo provvedimento venga criticato persino all'esterno e addirittura si ritenga possa essere inutile dal punto di vista tecnico. Ricordava come la Corte dei Conti abbia addirittura ritenuto poco credibili alcuni passaggi di questo DPEF. Ringrazio il Presidente per l'onestà intellettuale dimostrata nel volerlo rimarcare, nonostante fossero le sette di mattina, ma credo che questa sia anche una autodenuncia della pochezza di questo Documento. dicevo, siamo in presenza di un DPEF carente negli obiettivi e poco credibile nei numeri e nelle strategie per raggiungerli, un DPEF che dimostra tutta la debolezza dell'attuale maggioranza ed evidenzia tutte le contraddizioni che la caratterizzano.

ha perso il significato che aveva nel passato, quando, al di là dello stabilire l'indebitamento massimo, si indicavano anche le perimetrazioni, in modo che, poi, la finanziaria successiva non potesse che avere quelle linee direttrici. Così si stabilì nella legge di contabilità dello Stato, così finisce per non essere più, perché il Documento di programmazione

diceva Mann che "Il nuovo secolo sarà dominato dal danaro e dalla psicanalisi". Quale migliore occasione di un Documento di programmazione economico-finanziaria: di denaro se ne parla, di psicanalisi pure, quindi facciamo un po' di psicanalisi nei confronti del Governo e cerchiamo di capire qual è la reale

Il Governo, infatti, con un atteggiamento molto liberista, dice che non può favorire la crescita, se mai non può impedirla. Allora, se non posso impedirla, se debbo comportarmi come in Belgio e prendere le risorse per cercare di diminuire il debito pubblico, nel DPEF il Governo dice che lo farà attraverso pensioni, sanità e impiego pubblico.

Sulla sanità, vogliono mettere i *ticket*? Il vice ministro Visco questa mattina ha detto no, perché nella sanità c'è uno spreco assurdo. Vedete cosa fanno, li arrestano tutti, da Nord a Sud, dal Piemonte alla Sicilia, dalla Lombardia al Lazio e alla Puglia. A questo punto cosa vuole fare? Recuperare le spese della sanità con la Guardia di finanza? Mi sembra anche questo un programma che non esiste. Allora cosa resta? Resta l'impiego pubblico.

Signor Vice ministro, il Documento di programmazione economico-finanziaria, relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2007-2011 alla nostra attenzione, è di particolare importanza, perché delinea l'impegno programmatico del Governo di centro-sinistra per l'intera legislatura. Mi limiterò a due osservazioni: la prima riguarda il quadro complessivo della manovra prevista con la legge finanziaria del 2007. Gli obiettivi sono estremamente impegnativi, sia sul lato della finanza pubblica (dove si prevede, per gli anni 2007 e seguenti, una cospicua riduzione dell'indebitamento netto e un rilevante aumento dell'avanzo primario), sia sul lato dello sviluppo dell'economia e del perseguimento di una maggiore equità sociale. Per questo viene considerato necessario, nella prossima legge finanziaria, il reperimento di una somma notevolissima: 35 miliardi di euro. Nell'attuale situazione dell'economia si tratta di una somma quasi esorbitante. Personalmente, dubito che il reperimento di una tale somma sia effettivamente possibile. Ritengo, comunque, che non sarebbe saggio farlo. Nel caso che questo proposito venisse attuato, il suo effetto depressivo sarebbe grave. In effetti, lo stesso DPEF prevede che, per effetto della manovra in questione, lo sviluppo tendenziale del prodotto interno lordo si ridurrà nel 2007 dall'1,5 per cento all'1,2 per cento, il che non è certamente un fatto positivo, se si vuole promuovere l'economia. Il Documento non precisa nemmeno indicativamente come verranno reperiti questi 35 miliardi di euro, quanti saranno ottenuti tramite aumento delle entrate e quanti invece mediante il contenimento delle spese nei quattro grandi comparti della spesa pubblica Questa mancata precisazione, obiettivamente una carenza di trasparenza, non può non generare apprensione. La seconda osservazione riguarda le azioni previste a sostegno dello sviluppo del comparto delle imprese produttive. Al riguardo, va innanzitutto segnalata nel Documento la sostanziale contraddizione esistente tra il riconoscimento dell'importanza dell'obiettivo della crescita crescita e la mancanza di un'adeguata attenzione alla creazione delle condizioni che favoriscano l'investimento in capitale fisico ed umano da parte delle imprese e delle famiglie. In merito, basti ricordare varie disposizioni del provvedimento approvato qui ieri notte, relativo alla conversione in legge del decreto-legge Visco-Bersani, quali, ad esempio (e sottolineo ad esempio): le disposizioni fiscali retroattive, la sostanziale abolizione delle *stock options*, il cospicuo aumento degli obblighi burocratici da parte degli operatori economici, l'introduzione di vincoli di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, nonché il rafforzamento macroscopico dei poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Sono tutte disposizioni che tendono a disincentivare l'azione imprenditoriale, non certo a promuoverla. In complesso il Documento di programmazione economico-finanziaria analizza i problemi del comparto produttivo senza profondità e senza adeguato dettaglio. Le azioni di supporto prospettate, pur apprezzabili (come la promozione della concorrenza e la diminuzione del carico fiscale e contributivo) sono assolutamente insufficienti. Ne esaminerò ora le carenze più vistose. politica dell'energia, non viene fatta nessuna menzione dell'opzione nucleare. Ricordo al riguardo il proverbio latino: «*Perseverare est diabolicum*». E' dal novembre del 1987 che noi abbiamo colpevolmente abbandonato questa forma di energia primaria. Attualmente nel mondo il 16 per cento dell'energia elettrica è prodotto per via nucleare. In Europa tale percentuale sale al 35 per cento. Negli USA una ventina di grandi centrali nucleari progettate trenta anni fa hanno avuto recentemente l'autorizzazione ad una durata dell'esercizio di sessanta La tecnologia dei reattori nucleari ad acqua è ormai da considerare assolutamente sicura e provata. Il prezzo del petrolio ha raggiunto stabilmente i 70 dollari *per* *barrel*. L'Italia è un Paese che deve importare l'85 per cento del suo fabbisogno energetico. Non esiste attualmente né è prevedibile che venga messa a punto nei prossimi decenni alcuna altra tecnologia energetica di prestazioni paragonabili al nucleare. Nel Documento invece di parlare di nucleare si prevede un rilevante sviluppo delle agroenergie, è una barzelletta. Lasciatemi citare questi numeri. Con le coltivazione di colza o girasole si raggiungono rese dell'ordine di una tonnellata di biodiesel per ettaro e per anno. Nel 2005 il consumo interno di petrolio e prodotti petroliferi in Italia è stato di 86 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio. Se noi volessimo produrre un milione di questi 86 milioni mediante biodiesel dovremmo coltivare 1 milione di ettari, cioè 10.000 kmq, la superficie

Del carbone non si parla, ma del Protocollo di Kyoto sì. Osservo una sorta di sadomasochistico piacere nella sottolineatura presente nel Documento della grande rilevanza anche in termini di costo che avranno gli impegni previsti per l'Italia da questo Protocollo negli anni a venire. In sintesi, le azioni del Governo nel settore energetico previste dal Documento appaiono totalmente inadeguate rispetto alla drammatica esigenza propria del nostro Paese in questo settore. Gli interventi prospettati per favorire la concorrenza nel settore del gas, (tra cui si nota tra le righe l'intenzione di introdurre forme di separazione proprietaria tra le società fornitrici di gas e le società aventi possesso di reti di distribuzione e impianti di stoccaggio) sono oggettivamente di entità assai limitata. Politica delle infrastrutture. Nel Documento l'impegno del Governo per l'essenziale sviluppo dell'infrastrutturazione viaria e ferroviaria del Paese risulta molto generico, privo di precisi impegni, perciò niente affatto tranquillizzante. Anzi, in vari punti dell'intervento si prevedono «interventi correttivi» che rallenteranno cospicuamente i processi di infrastrutturazione avviati nella scorsa legislatura dal Governo Berlusconi. Tra questi segnaliamo per le inevitabili conseguenze dilatorie la promessa del ricorso alla via ordinaria per la valutazione dell'impatto ambientale del TAV in Val di Susa, la previsione di una grossa ristrutturazione dell'ANAS spa per adeguarne ruolo e funzione, nonché la previsione di una profonda revisione del sistema giuridico degli appalti pubblici. Signor Presidente, le chiedo di poter allegare agli atti la restante parte - per altro breve - del mio intervento.

Se ho capito bene, il senatore Baldassarri ha sostenuto che il Documento di programmazione economico‑finanziaria, in forza della legge n.

In buona sostanza, il senatore Baldassarri avrebbe richiesto che la tabella che questa mattina il Governo ha opportunamente fornito, quella del conto economico della pubblica amministrazione a sia accompagnata dal conto economico analitico, secondo questo stesso livello di analiticità, programmatico. vorrei in primo luogo affermare, con grande nettezza, che la legge n. 468 non prevede che il Documento di programmazione economico‑finanziario abbia questo contenuto. Sono andato a rivedermi per sicurezza l'articolo 3 della succitata legge che definisce, per ciò che riguarda il quadro programmatico, l'elenco delle informazioni che il DPEF deve fornire

;dobbiamo avere il rapporto tra volume globale del debito e prodotto interno lordo (e questo rapporto è previsto); dobbiamo avere i valori assoluti del disavanzo corrente del conto della pubblica amministrazione al netto degli interessi e al lordo degli interessi - e questo dato è deducibile dal quadro programmatico presentato all'interno del DPEF, per quanto, e questo è un limite, non analiticamente indicato - e poi dobbiamo avere, invece, sembrerebbe dedurre il senatore Baldassarri,

L'articolazione degli interventi correttivi però, signor Presidente, non è mai stata effettivamente definita pienamente in sede di Documento di programmazione economico-finanziaria, tanto è vero che sistematicamente, al momento della predisposizione della legge finanziaria, cioè della scelta dell'articolazione specifica degli interventi nel quadro degli obiettivi generali di finanza pubblica fissati dal DPEF, si ricorre alla presentazione della Nota d'aggiornamento. Prima della presentazione di questa nota d'aggiornamento, una tabella analitica dell'articolazione degli interventi è ovviamente non disponibile, non lo è quest'anno come non lo è stata

la risoluzione della minoranza, anche se non ho potuto esaminarla) che naturalmente, quando l'articolazione degli interventi sarà, essa sì, definita, nella fase immediatamente precedente la presentazione della legge finanziaria, una eventuale Nota d'aggiornamento del DPEF potrà contenere quel livello di informazioni che sono richieste dalla lettera f dell'articolo 3 della

*(Ulivo)*. Sto intervenendo nell'ambito dei minuti concessi al mio Gruppo, non sto rubando minuti a nessuno. Per quanto riguarda l'intervento sul merito, vorrei soffermarmi solo su un punto. Per uno Stato molto indebitato come il nostro, la credibilità è tutto, gli economisti la chiamano merito di credito; la trasparenza dei conti è un fattore fondamentale di credibilità e ha rilievo economico. Su questo punto, l'ultimo rapporto del Fondo monetario internazionale, a proposito dell'Italia, parla esplicitamente di conti opachi, di enorme rilievo - durante l'audizione sul Documento di programmazione economico-finanziaria, qualche giorno fa, alla Camera dei deputati, ha affermato testualmente che sono «oscuri» i «criteri che presiedono all'elaborazione del quadro a legislazione vigente», cioè quello di cui parlavo in in precedenza e che è stato fornito quest'anno con un livello di analiticità che non ha precedenti. Sono dunque oscuri i criteri, c'è chi trova modo di divertirsi di fronte a questo dato, ma io mi preoccupo, perché questo dato non è né di destra né di sinistra, è un problema del Paese. La trasparenza dei conti pubblici è un bene pubblico fondamentale, la credibilità del Paese, per uno Stato indebitato come il nostro, è uno dei fattori decisivi di una buona politica economica. Ora, a questo proposito vorrei far notare che se la Corte dei conti, il massimo organismo di controllo, sostiene che in generale sono oscuri i criteri con cui viene costruito il quadro tendenziale a legislazione vigente, è tutta la sessione di bilancio, che si fonda sul bilancio a legislazione vigente, vigente, a ricevere da questo giudizio un'ombra su se stessa molto forte. Lodevolmente il Governo, facendo qualcosa di cui non ho notizia di precedenti,

ad un rafforzamento e ad un mutamento delle caratteristiche del lavoro della Ragioneria generale dello Stato e, più in generale, del Ministero, che sia finalizzato a rendere i conti più trasparenti e affidabili di quanto non siano oggi. In particolare,si impegna a rendere disponibili per gli altri organi coinvolti nella decisione di bilancio questo livello di informazioni

impegna il Senato in un'attività di assoluto rilievo, che riguarda intanto il rafforzamento del Servizio del bilancio del Senato della Repubblica,

anche nel nostro Paese si costruisca qualcosa che somigli al centro parlamentare di controllo dei conti pubblici e di analisi dei conti pubblici più prestigioso del mondo: il Servizio del bilancio del Congresso americano.

oppure il tema della costruzione di un'Autorità indipendente si proporrà oggettivamente come l'unica soluzione possibile. La difesa della distinzione tra Senato e Camera su tale questione è un'operazione di retroguardia. Bisogna avere

che caratterizza il Servizio del bilancio del Congresso americano, mutando o cambiando ciò che si deve e considerando il diverso livello di organizzazione, di disponibilità di risorse proprie di queste due istituzioni parlamentari. Questa questione, apparentemente di carattere tecnico, ha un'enorme rilievo per la politica economica e di gestione della finanza pubblica dei prossimi anni, su cui mi sono permesso di richiamare l'attenzione di tutti voi. *(Applausi dai

Siamo all'avvio di una legislatura ed alla fase finale della discussione al Senato del primo Documento di programmazione economico-finanziaria. A me sembra che stiamo affrontando un problema, su cui è necessario trovare delle convergenze nelle analisi e possibilmente anche nelle soluzioni perché i problemi del Paese sono gravi, come abbiamo cercato di argomentare e di dimostrare.

Quando qualche collega ha parlato di un Documento di programmazione economico-finanziaria basato sulla sabbia, ha detto semplicemente una cosa non vera. Possiamo essere in dissenso rispetto alle soluzioni da adottare, ma dobbiamo riconoscere che i problemi indicati,

Se volete, andata a prendere quanto detto dal ministro dell'economia, Siniscalco, due anni fa: aveva già posto allora questa stessa questione. Si rileva l'esigenza quindi di riconoscere un punto di partenza ed una base di analisi. Faccio un altro esempio: qualcuno nell'intervento ha accusato il Documento di programmazione economico-finanziaria di introdurre tasse; ha contrapposto una strategia di riduzione del carico fiscale realizzata nei cinque anni precedenti ad una nuova strategia di imposizione di nuove tasse che avremmo in mente di fare. La polemica sulle tasse! Colleghi, nel 2006 la pressione fiscale - lo ha detto la Corte dei conti nelle audizioni - è tornata al livello del 2001. Non so se aumenteremo o ridurremo le tasse. Abbiamo intenzione di ridurle secondo la strategia indicata nel Documento. Non so se lo faremo. So per certo che nei cinque anni precedenti le tasse non sono state ridotte. Nel 2005 - ci ricorda sempre la Corte dei conti - la manovra aumenta la pressione fiscale sulle imprese per otto miliardi di euro. Non so cosa riusciremo a fare, se riusciremo a realizzare quanto ci siamo dati come programma. Penso di sì! So per certo che l'anno scorso le imprese sono state gravate per otto miliardi di euro in più di oneri sul fronte fiscale. Penso che la premessa Penso che la premessa per qualunque confronto che dobbiamo fare, a mio avviso, su questi problemi, sia riconoscere la realtà della situazione.

già detto dal collega Boccia questa mattina. A parti invertite abbiamo vissuto insieme lo stesso caso: negli anni precedenti è stata sempre consegnata alle Camere la Tabella del conto delle pubbliche amministrazioni negli andamenti programmatici. Prendiamo atto che questa volta non c'è. Veniamo al ragionamento sull'analisi e sulle indicazioni di politica economica, seguendo anche l'invito del collega Morgando appena ricordato. Un piccolo cenno fuori testo: il collega Mannino nel suo intervento - facendo capire un po' la situazione in Europa ha citato il caso di un'Europa che sta discutendo la dismissione di 400.000 ettari di vigna, in una logica di mercato chiuso europeo in cui, data la quantità prodotta di vino, si determina un eccesso di vino e quindi bisogna ridurre la terra coltivata. Abbiamo avuto casi simili, in passato, con le mucche, con il latte, con il burro e quant'altro. Ebbene, mentre l'Europa sta pensando di tagliare 400.000 ettari di vigna, c'è un programma in Cina per coltivare, nei prossimi cinque anni, quattro milioni di ettari a vite, per produrre vino e invadere il mondo con il vino cinese. È un piccolissimo, banale esempio

il risanamento è il 100 per cento dello sforzo che ne viene fuori. Questa potrebbe sembrare un'analisi tecnica, invece nasconde un preciso patto politico con un preciso blocco sociale: è la scelta di far prevalere gli equilibri finanziari e gli interessi della finanza sull'economia reale. È una scelta legittima, trasparente, ma per noi non condivisibile. La conferma di questo si ha nel ragionamento più volte fatto nelle settimane scorse, quando lo stesso Ministro dell'economia, ma che altri esponenti della maggioranza e commentatori esterni, hanno dichiarato che la situazione della finanza pubblica nel 2005 è più grave di quella del 2002. Nell'audizione che è stata svolta con il Ministro dell'economia, il Ministro dell'economia, egli ha chiarito il suo pensiero, esplicitando esattamente cosa intendeva; ha detto che intendeva riferirsi all'andamento del debito pubblico e dell'avanzo primario.

La dinamica di crescita del debito è assolutamente diversa. Ciò che è vero è che l'avanzo primario, portato al 6 per cento nel 1997 per entrare nell'euro, oggi è ridotto allo 0,5 tuttavia, era già diventato 3 per cento nel 2001; il centro-sinistra aveva già mangiato metà del suo risanamento finanziario nell'anno di grazia 2001. 2001. Proprio questo dimostra la scelta del mero equilibrio finanziario: l'avanzo primario garantisce soltanto la stabilità finanziaria lo si raggiunge spiega qual è la strategia di politica economica che c'è sotto. Cari colleghi, vi do una formula per portare l'avanzo primario al 6 per cento da lunedì mattina della prossima settimana, esattamente quella che fu usata

la si trova anche nei dati dello stesso DPEF. Infatti, a fronte di un percorso di riequilibrio della finanza pubblica in termini di *deficit* pubblico

a fine periodo, con tutto questo enorme sforzo, toccando sanità, pensioni, pubblico impiego ed enti locali, nel 2011, per cento contro un tendenziale di 1,4. Questo enorme sforzo di risanamento finanziario avrebbe come contropartita lo 0,3 per cento di crescita in più. Negli anni 2007‑2008 si compensano (quindi non c'è nessun effetto), meno crescita nel 2007, un po' più di crescita nel 2008. Il tasso di disoccupazione, che nella precedente legislatura è sceso dal 10,7 per scenderebbe in questa legislatura dal 7,5 al 6,7: 0,8 per cento in cinque anni, cioè poco più dello 0,15 per cento Il *deficit* pubblico e il debito avrebbero una strana, massiccia *overdose* di riequilibrio finanziario, perché non solo staremmo sotto il tre per cento l'anno prossimo cosa anche corretta - ma arriveremmo a zero nel 2011. Zero *deficit* pubblico. Il debito pubblico, che occorre stabilizzare in rapporto al PIL, verrebbe condotto sotto il 100 per cento. Non si capisce quale sia l'effetto mitico di questa soglia del 100 Ciò che conta nella stabilizzazione del debito è la stabilità del rapporto, non la velocità della sua discesa. La controprova microeconomica di questo patto palese è trasparente: con i grandi interessi della finanza, delle grandi banche, delle grandi assicurazioni e delle grandi imprese, in Italia e in Europa, è la scelta sul cuneo fiscale. Così fu fatto nella precedente legislatura a governo di centro‑sinistra, quando si introdusse la DIT e la SUPERDIT per le grandi imprese e l'IRAP per le piccole e medie imprese. Riguardo al cuneo fiscale, il Governo chiarisca se sta parlando della riduzione dei contributi sociali o della riduzione delle tasse a carico dei lavoratori.

sottile e subdola alleanza che sta dietro i suoi titoli, e che sarà sicuramente nelle linee della prossima finanziaria, mancano due temi e tre soggetti. primo tema è la pressione fiscale: viene ridotta o viene aumentata? Non c'è scritto nel DPEF e lo ha anche detto, molto onestamente, il collega Morando. Noi chiediamo che ci sia scritto che obiettivo strategico è la riduzione della pressione fiscale perché questa è la molla allo sviluppo. Altro discorso è come si spalma nell'equità sociale la pressione fiscale tra i vari soggetti. Il secondo grande assente è la questione degli ammortizzatori sociali; è vero, noi abbiamo introdotto flessibilità ma non c'è nessuna linea di quantificazione di quali ammortizzatori sociali dovranno essere introdotti a partire dalla prossima finanziaria. Riguardo ai tre soggetti mancanti, la famiglia; che ne è del quoziente familiare? E per le piccole e medie imprese? Che ne sarà dell'IRAP? È opportuno dare a grandi banche, grandi imprese, grandi assicurazioni 10 miliardi di euro col cuneo fiscale? O piuttosto è opportuno, magari, togliere dalla base imponibile dell'IRAP il costo del lavoro? Ultimo grande assente: il Sud,

la senatrice Valpiana, il senatore Paolo Brutti e, infine, il senatore Tibaldi. La senatrice Valpiana ha detto giustamente che in questo DPEF non c'è la politica dei due tempi. È vero, c'è la politica di un tempo solo: il risanamento finanziario, punto e basta. Il collega Brutti ha sostanzialmente riprodotto in parte le annotazioni che ho riferito e ha chiesto al Governo di riflettere su quanto è stato detto. Infine, il collega Tibaldi - vorrei dirlo perché eravamo in due o tre in Aula e forse non tutti potranno leggere rapidamente il resoconto

Dica il Governo se queste richieste del collega Tibaldi sono coerenti con il DPEF e se saranno inserite nella prossima finanziaria.

arrivati a questo punto della discussione che si è protratta per un'intera giornata, cercherò di essere breve e sintetico. Desidero innanzitutto ringraziare

Il senatore Baldassarri ha parlato questa mattina dei problemi economici internazionali, dei problemi dell'economia europea rispetto a quella americana, dei problemi

una sottolineatura: è evidente che la politica economica europea non è adeguata alla sfida globale. Ciò dipende essenzialmente dal fatto che l'Europa non è un soggetto politico e dal fatto che mentre ci sono una Banca centrale e una moneta unica, non c'è una politica fiscale comune.

quella che consente, per esempio, agli Stati Uniti di esercitare il loro ruolo di Paese titolare della moneta di riserva senza nessun contrappeso. Questo, colleghi, porta esattamente a uno dei punti di dissenso più evidenti che si sono manifestati tra centro-destra e centro-sinistra nella passata legislatura - e anche in questa - in relazione a quello che dovrebbe essere il ruolo dell'Italia, dell'Europa e dell'Italia in Europa: quindi, su una visione strettamente nazionalistica o, addirittura, provinciale o, invece, battersi per un ruolo diverso del nostro Paese in Europa. Europa. Non è un caso che questo sia un punto centrale della nostra strategia, indicata nel Documento di programmazione economico-finanziaria oggi in discussione. Ciò ha anche a che vedere con l'atteggiamento che possiamo avere verso altri fenomeni, perché è evidente che i Paesi emergenti creano un problema ai Paesi già sviluppati.

qui il senatore Mannino, che produce un ottimo passito. Penso che se il senatore Mannino e gli altri produttori come lui vendessero il loro prodotto in Cina,

di nicchia, caratterizzato da produzioni che sono, rispetto alla domanda globale, di nicchia e il suo problema quindi è migliorare la qualità e competere in modo da

ed ho l'impressione che questo significhi che non siamo consapevoli della realtà del nostro Paese, perché io dico che la situazione attuale è anche peggiore di quella del 1992,

Venezia, che era stata uno dei centri di potere del mondo per alcuni secoli, ad un certo punto perde la scommessa della modernizzazione per quel che riguarda l'evoluzione sia della navigazione (e quindi il passaggio alle navi a vela rispetto a quelle a remi) sia degli armamenti e comincia un lento declino. In quel periodo, i veneziani non stavano male, né soffrivano la fame, anzi continuavano a far feste e carnevali, finché un giorno arrivò Napoleone Bonaparte e, senza sparare un colpo di cannone, occupò la città e la storia si concluse. Se guardiamo i dati relativi al nostro Paese in Europa e rispetto a quel che succede altrove, notiamo una difficoltà vera

rigidità comportamentali, oltre che giuridiche ed economiche. Un Paese che ha bisogno di essere rimesso in movimento ed è su questo che il nuovo Governo si vuole cimentare: è questa la sfida. Anche quando si parla di riorganizzazione delle forze politiche, dietro vi è il problema di quale possa essere l'avvenire dell'Italia in questo secolo: ce la facciamo o siamo destinati ad una lenta consunzione? Bisogna cambiare. Quando indichiamo il problema della tutela del consumatore (altri possono parlare della concorrenza o delle liberalizzazioni), ci riferiamo ad un fatto di fondo, ad un fatto strategico. Non possiamo avere un Paese che vive di piccole corporazioni, di rendite, di protezione, né possiamo fare l'errore che è stato fatto nella scorsa legislatura, quando invece di affrontare tali questioni si individuò come questione principale quella della sconfitta del sindacato, pensando che fosse il sindacato la causa delle difficoltà di crescita del Paese. Non è così e lo vediamo tutti i giorni, e questo è un tema. è un tema. L'altro tema, pur affrontato nella manovra correttiva, è quello del comportamento fiscale degli italiani. Non è possibile che in Europa siamo il Paese con il livello di economia sommersa e di evasione fiscale più elevato: due volte quello degli altri Paesi.

un sistema che, oltre a essere poco concorrenziale, perché ovviamente l'evasione è concorrenza sleale, non è efficiente.

E questa è un'altra questione. Vogliamo risolvere qualche problema o semplicemente illuderci che si può andare avanti come per il passato? Vengo a un altro punto che è stato da molti sottolineato, da ultimo ancora dal collega Baldassarri, cioè al al risanamento separato dallo sviluppo e dall'equità. Ovviamente, non è così. Vedete, se gli equilibri finanziari non fossero importanti, nella passata legislatura avremmo dovuto avere un *boom* economico, ma nel momento in cui il disavanzo aumenta ed esplode e non si assiste a una crescita del reddito dovrebbe venire qualche dubbio

Ci dovremmo chiedere perché tutti i Paesi che vanno meglio hanno i conti in regola. Penso, allora, che il risanamento abbia molto a che fare con lo sviluppo.

ritengono eccessivamente contenute, da cosa derivano? Senatore Baldassarri, derivano dal fatto che non abbiamo voluto fare l'errore che avete fatto voi cinque anni fa. anni fa. Abbiamo voluto fare previsioni prudenti, perché se uno è prudente poi al massimo può avere buone sorprese, ma evita di trovarsi con una descrizione del mondo al 3 per cento di crescita composta l'anno e poi con un risultato di stagnazione o di recessione come quello che abbiamo sperimentato negli anni passati. negli anni passati. Quindi, penso che se avremo successo quelle cifre saranno più elevate e saremo ben lieti di aggiornarle e aumentarle.

che cosa sperimenta? Per prima cosa, un conflitto distributivo feroce tra chi è in grado di difendere il proprio potere di acquisto, o magari aumentarlo, e chi invece non è in grado di farlo. È quello che è avvenuto in Italia in questi anni. Dietro le variazioni dei prezzi si è celata un'enorme redistribuzione di reddito e di ricchezza;

consentitemi - le politiche tributarie fatte dal precedente Governo non sono state particolarmente orientate alla redistribuzione. Sappiamo perfettamente

Ciò significa che il finanziamento di quelle riduzioni avveniva attraverso recuperi di evasione, elusione e quant'altro. Una strategia del genere è assolutamente possibile. Naturalmente, questo non significa che possiamo - mi rivolgo anche ai colleghi di maggioranza che giustamente sono preoccupati

nel 2006 la spesa corrente primaria sarà cresciuta di due punti e mezzo di PIL e che le entrate tributarie si saranno ridotte di oltre un punto di PIL.

quattro. Non voglio ignorare il fatto che la crescita in questi anni è stata più bassa di quella potenziale,

non sono mai andato in televisione, né lo ha fatto il ministro Padoa-Schioppa, a fare denunce su buchi veri o presunti. Noi abbiamo effettuato una *due diligence* e i dati sono evidenti.

No, io parlo degli ultimi cinque, poi ci sono tutte le difficoltà che vengono da lontano e che noi non abbiamo mai negato, perché come stanno le cose lo lo sappiamo e non siamo persone che normalmente fanno demagogia. Quindi, la situazione oggi è tale per cui dobbiamo risanare adottando manovre strutturali. Non vi è più niente da tagliare in senso tradizionale; vi sono da modificare regole e comportamenti che hanno a che vedere anche con la spesa. Vorrei ricordare al senatore Ghigo, che questa mattina

Naturalmente, prendo atto della cortesia con cui vengono ascoltate le posizioni del Governo. Governo. Concludendo, signor Presidente, questa è la situazione del nostro Paese, questi sono i problemi. si prepara ad affrontarli nel modo più consapevole ed equilibrato, facendo pieno affidamento sulla sua maggioranza,

e sono anche consapevoli che nella passata legislatura non sono stati in grado di risolverli. Infatti, ciò che dicono alcuni di loro è semplice:

più impegnative e più utili per il Paese, ma - vivaddio! - in un regime democratico comanda la maggioranza e noi la maggioranza l'abbiamo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con i colleghi Maccanico e Villone - altri consensi però si sono aggiunti, da ultimo quello del senatore Biondi abbiamo presentato un emendamento aggiuntivo alla risoluzione sul Documento in oggetto, che ha come tema la riduzione dei costi della politica. Io sono favorevole a votazioni *bipartisan*, ma non mi è piaciuta molto la votazione *bipartisan* di ieri, quando molti di noi hanno intuito, da un balletto di precisazioni finali, che c'era stato un accordo unanime

Quanto al provvedimento di ieri, lo leggeremo e lo studieremo perché conosco la sua precisione. Comunque, nel momento cui si chiede al Paese una stretta dei consumi, credo che il sistema politico debba dare il suo contributo. Questo è il significato dell'emendamento che abbiamo presentato e che prego i colleghi di leggere e valutare; questa questa riduzione è essenziale, a mio avviso, per recuperare il rapporto di credibilità del sistema politico con il Paese, per recuperare la competitività del sistema Italia, per sfoltire il sistema pubblico da incarichi, competenze, società miste, società per azioni, relativi collegi e consigli di amministrazione, per fissare criteri rigorosi e trasparenti per la spesa pubblica e per le retribuzioni e i compensi di tutti coloro che vivono a carico della politica. Questo è il senso dell'emendamento. Se la riformulazione accoglie questi concetti, naturalmente, non ho nessuna difficoltà ad aderirvi. *(Applausi dal Gruppo FI e del senatore presentato dal senatore Salvi è la seguente: si mantengono i primi due punti della premessa: «una strategia efficace di contenimento della spesa pubblica non può prescindere della riduzione dei costi impropri della politica. Tale riduzione è anche un elemento essenziale per il recupero di competitività del Paese, su cui grava il peso di un sistema politico pervasivo e di un rapporto non corretto tra politica e amministrazione. altre parti dell'emendamento - affrontare numerosi problemi: gli oneri derivanti dal costo della politica, individuando con criteri rigorosi i soggetti che ne hanno diritto; diritto; la riduzione del numero degli eletti e il ripristino del carattere volontario della partecipazione politica e amministrativa; la semplificazione istituzionale, fermando ogni ulteriore incremento degli enti di rappresentanza territoriale e delle amministrazioni parallele.

delle esigenze sia di carattere contenutistico che sistematico. A me pare che con questa impostazione si possano risolvere entrambi i problemi. Preannuncio, qualora

al ripristino del carattere volontario della partecipazione politica e amministrativa. PRESIDENTE. Ho qualche perplessità sull'ammissibilità della riduzione del numero degli eletti in un Documento di programmazione economico-finanziaria. Senatore Salvi, la prego se capiscono il tipo di problema, può interessare anche a loro) "Condizionare il finanziamento pubblico ai partiti all'adozione di regole di democrazia interna, sulla base di norme e di leggi da adottare in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione".

perché, come previsto dal Regolamento, vi sia un filtro di ammissibilità. Trattandosi di una risoluzione sul Documento di programmazione economico-finanziaria, la lettura degli emendamenti consentirà ai Gruppi e ai singoli senatori di decidere come votare, ma consentirà anche alla Presidenza di vagliare il contenuto degli stessi. Pertanto, signor Presidente, nel lasso di tempo delle dichiarazioni di voto o se ritiene, attraverso

mi riservo di giudicare dell'ammissibilità perché non è specificato a quale categoria ci si riferisce. Ho suggerito, facendo una domanda, anche la risoluzione del problema, non la si vuole cogliere

preoccupazione che lei aveva espresso in ordine all'ammissibilità dell'emendamento relativo - diciamo così -ai costi della politica. Ho effettuato qualche verifica e qualche approfondimento anche sulla sovrapposizione del contenuto dell'altro emendamento, relativo al Mezzogiorno, con alcuni contenuti della risoluzione che metterebbero i due testi in contraddizione.

Sento che, anche se per motivi che non mi sono personalmente chiarissimi, il relatore e il Governo hanno espresso parere contrario. Quindi, d'intesa con gli altri presentatori, i senatori Maccanico e Villone, ritiro l'emendamento 2.2, auspicando un rapido approfondimento di temi - a mio avviso - importantissimi per la democrazia e il sistema politico italiano.

posto. Verrà comunicato in altra sede che le segnalazioni potranno essere fatte solo dai Capigruppo alla Presidenza e ai senatori segretari. Dichiaro chiusa la votazione. **Il Senato non approva.** *(v. Allegato

indicare il primo firmatario degli emendamenti, perché in questo contesto l'Aula, o almeno alcuni senatori, non hanno compreso di quale emendamento si trattava.

credo di dover supportare la valutazione e la considerazione del senatore Procacci. Io stesso su quell'emendamento, che non è di poco conto - anzi di forte significato politico - non ho avuto la percezione che lo stessimo votando.

Signor Presidente, onorevoli senatori, il Documento di programmazione economico-finanziaria rileva le difficoltà del nostro sistema Vorrei pregare il Presidente di assicurare il regolare svolgimento dei lavori. Dicevo, il Documento di programmazione economico-finanziaria rileva le difficoltà del nostro sistema del Paese: il calo della produttività totale, dei fattori della competitività, le difficoltà dei nostri conti pubblici, l'aumento delle disparità sociali. Dopo un esame realizzato con grande onestà intellettuale, il Documento passa a realizzare un'anticipazione che, per forza di cose, non può che essere molto generale e sommaria, delle previsioni normative che verranno messe in atto dal Governo in sede di manovra finanziaria per il 2007. L'importo della manovra che si dovrà realizzare, pari a circa 35 miliardi di euro, la contraddistingue come una delle strategie di bilancio più imponenti degli ultimi anni, seconda solo a quella del Governo Amato del 1992. Il Documento realizza una previsione che andrà ad incidere sui conti pubblici in misura pari al 2,3 per cento del prodotto interno lordo. Come sappiamo, una parte dell'intervento sarà riservata alla copertura del debito pubblico, una parte sarà riservata allo sviluppo del Paese. La prima condizione è strettamente legata alla seconda, in quanto non ci può essere sviluppo duraturo del Paese senza una seria politica di risanamento dei conti pubblici. La cosa evidente, messa in luce sin dalla presentazione del primo intervento di finanza pubblica attuato con il cosiddetto decreto Bersani, è che il Governo intende proporre solo interventi strutturali. Spariscono cioè le misure *one-off*, versione moderna delle cosiddette *una* *tantum* di antica memoria. Queste erano misure cuscinetto, che duravano l'arco di tempo in cui sviluppavano la propria azione e che servivano solamente a tamponare situazioni di bilancio orientativamente, ci aspetta un periodo che sicuramente - temo - non sia inferiore all'ora, quindi chi vuol lasciare l'Aula e consentire le dichiarazioni di voto darà prova di buona volontà. CUSUMANO *(Misto-Pop-Udeur)*. Nelle previsioni economico-finanziarie del Governo Prodi, non ci sono più - e non ci saranno scudi fiscali, condoni edilizi o fiscali. Si va ora verso l'allargamento della base imponibile, allo scopo di includere tra i contribuenti onesti quei soggetti che ora, grazie a leggi poco accorte e a sistemi di controllo inefficaci, hanno potuto godere di una sorta di impunità nell'elusione e nell'evasione fiscale. Proprio il recupero di base imponibile, il monitoraggio completo della spesa pubblica e il taglio degli sprechi e delle inefficienze nella pubblica amministrazione possono concorrere alla riduzione del debito pubblico e alla crescita del prodotto interno

Con queste premesse si possono definire le linee di azione che vedranno l'appoggio della nostra parte politica anche a un intervento mirato, intelligente e duraturo nei quattro grandi comparti della spesa pubblica. La prevista redistribuzione del carico fiscale deve però tenere conto della circostanza che le famiglie italiane sono le più penalizzate d'Europa. Gli effetti di quei pure minuti vantaggi che le famiglie italiane hanno ottenuto, prima con il raddoppio delle detrazioni e poi attraverso l'introduzione delle deduzioni per i familiari a carico con il secondo modulo fiscale devono essere mantenuti. Non vedrebbe il nostro appoggio un'abrogazione *tout court* del secondo modulo fiscale che non salvaguardasse i vantaggi in essere per le famiglie italiane. Né potremmo accettare una stratificazione dei redditi da Paesi socialisti, che non tenesse conto della presenza nella società del ruolo dei nuclei familiari e della esigenza dei giovani di costituirsi in famiglia (quella di diritto), di fare figli e di acquistare la loro prima casa.. Tutte queste esigenze hanno dei costi di cui lo Stato deve farsi carico e di cui la manovra finanziaria per il 2007 dovrà tenere conto. Siamo lo Stato in Europa che investe meno nella famiglia, il confronto con la Francia e con i quozienti familiari è quello cui dobbiamo tendere, ma non possiamo dimenticare che altri Paesi possiedono legislazioni estremamente premiali nei confronti della famiglia. Accanto al problema che riguarda la famiglia di diritto, si pone quello degli anziani. L'altro argomento fondante della politica dei Popolari-Udeur è il Mezzogiorno. Il processo di riforma degli aiuti alle aree depresse introdotto negli ultimi anni ha avuto l'enorme pregio di ridurre gli sprechi e le attribuzioni indebite di risorse.

le potenzialità delle imprese e attribuire loro finanziamenti a tasso agevolato e in conto capitale. Bisogna quindi proseguire con quegli strumenti, quali i contratti di programma, i patti territoriali, i contratti di localizzazione e i contratti d'area, in due parole con la programmazione negoziata, che ha dato finora buoni risultati nei piani di intervento per il Sud. Sono certamente fondamentali i requisiti di innovazione e competitività che devono possedere le imprese che usufruiscono di aiuti, ma lo Stato deve investire con maggiore coraggio nelle infrastrutture del Mezzogiorno. C'è ancora una differenza troppo accentuata tra il sistema infrastrutturale del Sud e quello del resto del Paese. Tale dissonanza aumenta se consideriamo che tra le infrastrutture necessarie allo sviluppo ci sono quelle della ICT. Il divario creato con il *gap* tecnologico tra Nord e Sud, deve essere in tempi rapidi abbattuto: ne va di mezzo lo sviluppo del Mezzogiorno e dell'intero Paese. Per quanto riguarda l'agricoltura e la pesca, ci aspettiamo che vengano confermate le misure di vantaggio fiscale e contributivo già in atto in questi settori che stanno affrontando una generale ristrutturazione del quadro degli aiuti in sede europea. Insomma, chiediamo una manovra finanziaria equilibrata, che premi le famiglie e che affermi un'attenzione concreta per il Mezzogiorno. Confidiamo in un ascolto attento delle nostre istanze da parte del Governo e del Ministro dell'economia ed esprimiamo il voto favorevole del Gruppo Misto-Popolari-Udeur alla risoluzione del centro-sinistra

una cornice programmatica entro la quale si collocherà o dovrebbe collocarsi l'attività dell'Esecutivo nei mesi a venire, è evidente che da esso è possibile intravedere la filosofia generale di un Governo che ha preteso sin dai primi giorni di definirsi come un Governo di svolta. Salvo poi, come nel caso delle liberalizzazioni, fare non svolte ma giravolte ai primi ostacoli. Figuriamoci se dai tassisti si dovesse passare ai grandi poteri dei settori strategici. Ciò premesso, dichiaro da subito il mio scetticismo sulla capacità di questo Esecutivo di affrontare i grandi temi e i grandi obiettivi che con enfasi il DPEF consegna alla nostra attenzione. Tra questi temi e grandi obiettivi è, come da tradizione, assente il Mezzogiorno, e non solo, o non tanto, per insufficienza di risorse, quanto per cultura consolidata di un ceto dirigente da sempre abituato a trattare il Sud, anche per colpa dei meridionali, come argomento residuale a cui destinare modeste risorse, utili, forse, per un modello tardo-assistenziale ma assolutamente inadeguate per assicurare una pur modesta inversione dei percorsi di crescita. Quel che è accaduto qualche minuto fa è emblematico del disinteresse, oltre che della Presidenza,

lasciati soli, abbandonati, senza un supporto, quando in quest'Aula ci sono grandi solidarietà, anche molto rumorose! *(Applausi del Certo, si tratta di una coerente e rigorosa analisi del quadro economico del Paese. Non si indulge, come è avvenuto qualche volta, ad un ottimismo di facciata, né si ipotizzano flussi finanziari in entrata buoni, forse, per effetti placebo incompatibili con i vincoli internazionali entro i quali siamo collocati. Inoltre, il quadro descritto appare impietoso su un tema che dovrebbe condurre a più attenta riflessione anche le rappresentanze associative di quel mondo dell'impresa troppo spesso impegnate a giudicare con scarsa indulgenza e qualche volta con sospetta faziosità i limiti e le carenze del sistema politico del nostro Paese. Mi riferisco al dato sulla produttività e al ruolo che in questo campo dovrebbe essere svolto dagli attori principali dello sviluppo, gli imprenditori. Non vi è dubbio che la produttività non è il semplice frutto dell'intrapresa, esso è certamente la conseguenza di un insieme complesso di variabili: dalle infrastrutture alle relazioni industriali, dal clima politico ai processi di innovazione; ma se guardiamo al dato e, soprattutto alle date che segnano il declino, colpisce la coincidenza con le manovre finanziarie e con il clima complessivo che ha accompagnato l'ingresso dell'Italia nell'area dell'euro. È come se questo evento, che avrebbe dovuto chiamare tutti a maggiore responsabilità, avesse invece deresponsabilizzato 1'insieme degli attori dello sviluppo. E sarà bene che su questo tema il Governo intervenga seriamente, legando trasferimenti e politiche di incentivazione ai soggetti più responsabili, che facciano del legame produttività-competitivita il cardine della loro attività. Certo, un drenaggio di 35 miliardi di euro, dei quali 15 da destinare allo sviluppo e alla crescita, è una vera terapia d'urto; personalmente ritengo che potrà avere effetti limitati dal lato della domanda se si agirà, come pare, soprattutto su quella vasta area di reddito che sfugge alla responsabilità della democratica partecipazione agli oneri di governo di un Paese moderno. Evito volutamente di utilizzare il termine «evasione», che richiama non solo penosi fallimenti, oltre che sgradevoli complicità diffuse, ma in quanto evoca una cultura della sinistra statalista che interpreta l'intervento pubblico quasi esclusivamente in termini punitivi e non propositivi. Certo, che le liberalizzazioni annunciate e i recuperi auspicati non potranno avere effetti risolutivi nel breve periodo, mentre è al contempo evidente che eventuali disattenzioni o erronee valutazioni sui settori e sui redditi sui quali trasferire l'onere della manovra, potrebbero avere ricadute pesanti sulla domanda con effetti improvvidi sulla fragile e anemica ripresina in atto, trainata più dal quadro internazionale che da effettiva dinamizzazione delle variabili interne. Capitolo a parte merita il comparto pensionistico. L'idea che ogni intervento debba passare da un processo di condivisione è certamente corretto, ma è altrettanto noto che nel nostro Paese la concertazione rischia di avere esiti, alle volte, persino paradossali: anche in questo caso separato il privilegio dal bisogno, evitando di tutelare il primo non potendosi poi, ovviamente, non tutelare il secondo (quantomeno speriamo). Il sistema pensionistico va, dunque, ridisegnato senza atteggiamenti punitivi, ma evitando che frange parlamentari, più che sindacali, definiscano sistemi di relazione lobbistici a danno del Paese. Per quanto attiene alle infrastrutture, si definiscano una volta per tutte le priorità strategiche per lo sviluppo del Paese, evitando il sistema dei veti e dei ricatti incrociati, e superando, per favore, questo imbarazzante documento costituito dall'allegato infrastrutture al DPEF, che ha messo in estrema difficoltà la stessa maggioranza in Commissione, costringendola ad esprimere un parere, frutto di faticose mediazioni, nel quale si palesano critiche rilevanti per i limiti evidenti del documento governativo. Dico questo perché voglio capire se i silenzi, ad esempio, sul ponte di Messina sono la conseguenza di una strategia seria sulle priorità infrastrutturali del Paese, ed allora vogliamo comprendere e studiare i contenuti di tale strategia anche in termini di asse dello sviluppo, o al contrario, siccome il Ponte era una priorità del Governo di centro-destra, ed è stato giudicato quasi un'opera di regime, necessariamente il centro-sinistra deve contrastarlo, quasi ideologicamente, anche sotto la spinta di un ambientalismo miope e di maniera, che non si occupa invece, per esempio, del drammatico inquinamento provocato dalle devastanti raffinerie insediate in Sicilia in alcuni dei litorali più affascinanti dal punto di vista paesaggistico. E veniamo dunque al tema del Mezzogiorno. La supponenza con le quali viene affrontato il tema nel DPEF è indicativo di una cultura politica diffusa che guarda al Sud come un peso ed un fardello del quale occuparsi quasi solo per dovere istituzionale. In questo Documento non si sono salvate nemmeno le apparenze: è trattato nell'ultima pagina con i contenuti di un compitino da ripetente senza pudore. Dunque, filiera agro-alimentare, turismo culturale alla Goethe e rivisitazione dei sistemi urbani sono i generici compiti assegnati al Sud. Ciò che ci mortifica è l'attento sforzo di evitare qualsiasi impegno programmatico. La totale assenza di una strategia che comprenda il ruolo del Sud e della Sicilia nell'area mediterranea, quando preme alle porte l'area di libero scambio che può trasformarsi, se non guidata politicamente, da grande opportunità in nuova, drammatica congiuntura economica e sociale. La superficialità con la quale si evita di affrontare il tema dei processi di incentivazione mirati ad invertire tendenze di crescita anchilosate dallo scadente sistema delle infrastrutture esistenti è insopportabile: la gravissima carenza di opere che penalizza il Mezzogiorno, e che viene costantemente accertata da qualsiasi onesta rilevazione statistica sulla dotazione infrastrutturale complessiva del Paese, non è indicata in questo DPEF nemmeno tra gli *handicap* primari per lo sviluppo. Ci si spieghi perché sulle infrastrutture si elenca una graduatoria tra opere appaltate, progettate e non appaltate, o da progettare, ed il Ponte è comunque assente, pur essendo appaltato e dotato di una quota di finanziamento importante, con la grave probabilità di incorrere in responsabilità economico-patrimoniali a carico dell'Erario, considerati gli obblighi contrattuali ed i vincoli di destinazione che assistono le risorse appostate in Fintecna a tale scopo, le uniche, tra l'altro - e questo è veramente paradossale - attraverso cui si ritiene di finanziare un nuovo, ipotetico ed indefinito piano di investimenti per il Mezzogiorno. Così l'assenza di un qualsiasi riferimento concreto, men che meno di un vero piano infrastrutturale, non è casuale, né conseguenza del conflitto eco-ambientalista; molto più semplicemente non c'è, perché il Sud non riveste alcuna valenza per le strategie di sviluppo del Paese, che, dopo aver puntato da sempre su altri territori, dovrebbe pur spiegare le ragioni vere degli attuali indici di produttività, della scarsa competitività internazionale e di una delocalizzazione dell'apparato produttivo che sul «piccolo è bello» aveva costruito il mito di un sistema Italia deludentemente fragile e pieno di contraddizioni. si spieghi perché si dice no (il silenzio del DPEF è più fragoroso di un netto rifiuto) alla fiscalità di vantaggio, e non si dice sì neanche ad un cuneo fiscale sul costo del lavoro applicato in modo differenziato per favorire nuovi investimenti al Sud, con il rischio evidente che venga applicata, invece, una normativa indistinta tutto il territorio nazionale che produrrebbe effetti gravissimi sulla economia delle aree sottoutilizzate. Il Sud ha smesso da tempo il rivendicazionismo volgare e di facciata, magari solo nelle sue espressioni politiche più responsabili, e chi come noi oggi parla di autonomia, lo fa chiamando in causa, nella responsabilità del dissesto, soprattutto le rappresentanze senza delega di tanto ceto politico meridionale. Almeno per l'attenzione che si deve a questa cultura politica da un Governo che vuole essere di svolta, pretendiamo il rispetto del valore del dialogo anche su elementi di dissenso, non questa superficiale supponenza per territori d'oltremare.

realistico nei dati e nelle analisi, un Documento che traccia il quadro di un Paese reale che deve affrontare molte difficoltà, ma che vuole affrontarle con uno spirito unitario e ce la può fare. La nostra risoluzione, inoltre, uno sforzo in più. Lo sforzo, cioè, di volgere lo sguardo dalle analisi macroeconomiche, dai numeri, dai dati, alle persone, ai soggetti, a quelle persone cioè che nella fattibilità e nelle prove di fattibilità di questo documento porranno le loro speranze, la loro vita. Si tratta di milioni di persone, innanzitutto, degli *outsider* attuali, giovani che cercano più elevati livelli di qualificazione e sbocchi professionali certi; delle donne che cercano in un *Welfare* rinnovato e riqualificato la compatibilità della loro doppia presenza, nel lavoro e nella famiglia; dei molti lavoratori anziani che non intendono sciupare, buttar via una vita di lavoro ed essere costretti a una precoce mobilità, ad un precoce e non voluto pensionamento -

Si tratta, cioè, dei cittadini del nuovo secolo con il loro antico desiderio di realizzazione personale e di sicurezza. i desideri di realizzazione personale e di sicurezza vanno coniugati con le nuove compatibilità, con un nuovo *Welfare*, con la sfida dell'elevamento dei fattori di produttività globale.

Visco che non c'è più nulla da tagliare ma tutto da modificare, tutto da ristrutturare. Sappiamo che questa strada avrà le sue asprezze. La nostra risoluzione, inoltre, lavora di fino; guarda al Mezzogiorno per il quale ha definito, ha estrapolato uno specifico capitolo, una specifica riflessione, una specifica azione propositiva e guarda anche, se proprio si vuole andare nel dettaglio, alle zone disagiate di montagna, di cui si è parlato nel dibattito, chiedendo il rifinanziamento del Fondo per la montagna. Non dimentichiamo infatti che nella montagna italiana, dal Nord al Sud, 70 per cento dei piccoli comuni laddove si stringe il vivere civile; zone di emarginazione, ma anche di nuove risorse, di nuove speranze, di compatibilità nuove, di tutela del territorio. La nostra risoluzione si impegna, inoltre, per la trasparenza dei conti pubblici e guarda con sensibilità alla ricaduta nella società civile dei provvedimenti economici che vuole mettere in campo: si pensi alle parti importanti sulla emigrazione o, ancora, all'elenco di quelle riforme che non costano, come la semplificazione amministrativa e la tutela dell'infanzia, che vanno fatte. Si pensi alla dimensione di internazionalizzazione delle imprese, una dimensione nuova, che va guadagnata, e presto, con convinzione, in una corsa contro il tempo. Il Gruppo Per le Autonomie, quindi, voterà con convinzione la mozione che ha anche contribuito a stendere, perché ci piace pensare che in questa mozione sono contenute le sfide del futuro, perché è esattamente al futuro che guarda con impegno e, appunto, con senso della sfida.

diversità di questo Documento di programmazione economico-finanziaria rispetto a quello presentato nel 2001 e rispetto a tutte le manovre precedenti, per analisi, scenari e obiettivi.

il punto di arrivo e un passo in avanti. Il DPEF è caratterizzato, innanzitutto, da una grande sfida: quella di poter coniugare rilancio economico, risanamento, equità, redistribuzione del reddito e politiche sociali. Nessuna politica dei due tempi: è stato detto chiaramente nel DPEF e ancora più chiaramente nella risoluzione che stiamo per votare. votare. Il risanamento, lo sviluppo sostenibile e l'equità, infatti, devono procedere di pari passo, perché non vi potrà essere risanamento se non sarà supportato da forti politiche di sostenibilità sociale e ambientale.

per la manovra di rientro, per realizzare un approccio più morbido e diluito sul fronte della riduzione della spesa pubblica, avendo, quindi, più risorse per le politiche sociali, territoriali e di rilancio dell'economia. tuttavia, è stata accolta e si è concretizzata nella risoluzione, con l'impegno del Governo a valutare con più precisione il percorso di rientro, in relazione al profilo temporale degli effetti strutturali delle misure.

si evidenzia la necessità dell'uso di indicatori ambientali e sociali da affiancare ai tradizionali indicatori macroeconomici. Nella risoluzione tale indicazione si rafforza ed è più chiara. Un'analisi di questo tipo è già presente nel DPEF, sul fronte degli indicatori della povertà e dell'istruzione. Proprio dall'analisi degli indicatori della povertà

attraverso l'introduzione dei parametri della qualità sociale e ambientale, per cominciare concretamente a scommettere su una politica economica e finanziaria nuova, che non abbia più solo il mercato

che questa idea di crescita possa evolvere sempre più verso uno sviluppo sostenibile ed equo. In questo DPEF e nella risoluzione si cominciano a delineare

qualifica la tutela ambientale come componente essenziale per la competitività del Paese, e finalmente integra l'ambiente nell'economia, in tutti i suoi settori. Non solo si fa riferimento all'applicazione del Protocollo di Kyoto ma, proprio nella risoluzione, si indica la strada delle forti iniziative di carattere strutturale per raggiungere gli obiettivi di Kyoto, inserendo tra queste diverse politiche pubbliche e puntando decisamente sulle fonti rinnovabili, con incentivi e senza tetti di produzione.

economia, a cui faceva riferimento anche il vice ministro Visco nella sua replica, si annette sul fronte del sistema agricolo e del sistema agroalimentare più in generale, un grande valore strategico proprio per la competitività e per uno sviluppo basato sulla qualità, sulla distintività e quindi sulle risorse, ai valori e alle eccellenze dei nostri territori. Turismo e cultura come volano, finalmente insieme, per una nuova economia che coniughi salvaguardia e valorizzazione dell'enorme patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Qualcuno ha cominciato a parlare della carta delle qualità. Credo che questa sia una strada interessante su cui dobbiamo puntare sempre di più. Un Paese come il nostro o punta sulla qualità del sistema, sulla qualità e l'innovazione della produzione, oppure ha difficoltà a riprendere un percorso forte di rilancio. È importante ciò che è scritto nella risoluzione per quanto riguarda il superamento della legge obiettivo e della sua logica, tanto ridondante e faraonica, quanto inconcludente, per arrivare a un piano di opere pubbliche che sia imperniato sulla programmazione integrata del Piano generale dei trasporti e della logistica, e tesa a privilegiare la mobilità sostenibile e le opere utili, progettate con i territori e con la popolazione, e finalmente sottoposte a valutazioni di impatto ambientale. Si indica nella risoluzione la sospensione dell'*iter* di realizzazione del Ponte sullo Stretto per drenare risorse sulla rete ferroviaria, stradale e portuale del Mezzogiorno. Vorrei anche esplicitare le mie preoccupazioni in riferimento alla manovra, per quanto riguarda il lato della spesa sui quattro grandi comparti: il pubblico impiego, la previdenza, la sanità e la finanza territoriale.

sul reddito minimo di inserimento, sulla lotta al precariato, sulla riqualificazione del pubblico impiego, sul rilancio della politica abitativa. È una sfida che abbiamo davanti a noi, una sfida grande. È possibile conciliare quindi risanamento, politiche sociali, di equità e nuova qualità sociale e ambientale per lo sviluppo? Noi pensiamo di sì. Crediamo che su questo fronte, e pensiamo anche alla lotta all'evasione e ad una nuova politica fiscale equa, stiamo andando nella giusta Ce lo chiedono i cittadini; questo si aspettano i cittadini da noi per ritornare ad avere una speranza nel proprio futuro e in quello del nostro Paese.

una diatriba abbastanza evidente all'interno della maggioranza mi permette di svolgere considerazioni sulla chiusura del vice ministro Visco, il quale aveva detto pochi minuti prima «noi siamo la maggioranza e quindi comanderemo, governeremo»,

alle società di gestione immobiliare che hanno perso, a seguito della norma sull'indetraibilità dell'IVA, più di un miliardo di euro in Borsa, norma poi nel maxiemendamento che è stato approvato con la fiducia al Governo) un'ulteriore conferma. Mi sembra che si stia cercando di seminare vento, e chi continuerà a farlo penso che non potrà che raccogliere tempesta. *(Applausi

Questo DPEF, però, non piace neanche a Verdi e Comunisti Italiani e non piace soprattutto alla CGIL, alla CISL e alla UIL. Secondo il Ministro Ferrero e tutta Rifondazione Comunista, perché si prefigurano tagli alla spesa sociale, secondo le organizzazioni sindacali, invece, perché i tagli alla spesa, quindi anche alla spesa sociale, non sono stati concertati. Anche il rialzo all' inflazione programmata dall'1,9 al 2 per cento richiesto dai sindacati, è stato deciso dal Governo in autonomia, senza alcuna negoziazione. Abbiamo un DPEF che annuncia una riduzione di debito pubblico in cinque anni di otto punti, pari a 120 miliardi euro ossia 230.000 miliardi di vecchie lire, ma non dice come; perché se lo dicesse, il giorno dopo la sinistra antagonista uscirebbe dal Governo. Anche noi leggendo le 175 pagine del documento in esame, non abbiamo capito come dovrebbe avvenire il risanamento dei conti pubblici con un avanzo primario ipotizzato al 4 per cento e una bassa crescita. Senza l'aiuto della fantasia, questi risultati si possono ottenere solo con un aumento delle entrate e una forte riduzione delle spese. Il Governo ha indicato che si muoverà su tre fronti: crescita, risanamento ed equità. Crescita e risanamento dovranno sostenersi reciprocamente, l'equità sociale e fiscale dovrà essere il parametro di riferimento delle misure d'intervento. Come hanno detto il ministro Ferrero e i sindacati, il documento in discussione lascia intravedere il risanamento prima della crescita, quindi una politica dei due tempi su quella della contestualità. Reddito di ultima istanza, fondo per i non autosufficienti, recupero del *fiscal drag*, innalzamento delle pensioni minime, restituzione dell'imposta negativa per gli incapienti, che sono stati i temi forti della campagna elettorale di Bertinotti e Diliberto, che hanno dato la legittimazione elettorale a questo Governo, sono spariti dall'agenda politica di questo Governo e di questo DPEF. Non fanno parte di quelle politiche positive per la promozione sociale dei singoli e della famiglia, anzi sulle politiche sociali a sostegno della famiglia si torna indietro rispetto alle conquiste fatte dall'odiato Governo Berlusconi. Il DPEF, partendo dal contesto internazionale, riconosce che il problema dell'economia italiana è quello della scarsa produttività: il costo di un prodotto in Italia è superiore a quello di altri Paesi per lo stesso prodotto. Questo peso riduce la nostra competitività nel commercio internazionale. Il documento riconosce che questo problema ha radici profonde, che va oltre la congiuntura sfavorevole degli ultimi anni; non è dunque colpa del Governo Berlusconi. L'euro ha dato maggiore stabilità finanziaria al nostro Paese, ma ha evidenziato la debolezza del nostro apparato pubblico e i ritardi di ammodernamento del nostro sistema produttivo. La globalizzazione da una parte e l'invecchiamento della popolazione italiana dall'altra, con il saldo naturale negativo, ha drammatizzato le politiche di intervento, rendendole improcrastinabili. L'economia mondiale nel 2005 è cresciuta del 4,7 per cento, quella degli Stati Uniti dell'1,7, dell'Europa dell'1,3, dell'Italia dello 0,6 per cento: mentre tutti corrono, noi passeggiamo. Il 2006 mantiene questo *trend* di crescita con maggior fortuna per l'Europa e l'Italia, ma per il 2007 si prevede un rallentamento. Materie prime e petrolio sono cresciuti a ritmi preoccupanti per un Paese trasformatore come l'Italia. Il prezzo del petrolio, da 38 dollari a barile del 2004 è passato a 55 dollari nel 2005, a 70 nel 2006 e si prevede che superi gli 80 nel 2007. Le tensioni geopolitiche nell'area dei maggiori produttori di greggio non fanno presagire nulla di buono, visto che la crisi, è crisi da offerta. Altro dato che ci fa pensare è la riduzione della domanda interna della Germania, causata dalle politiche di rientro del *deficit* della Merkel. La Germania è uno dei maggiori partner commerciali del nostro Paese. Altra considerazione che ci dovrebbe far pensare è riferita ai determinanti della buona crescita del 2006: +1,5 per dovuta a fattori non ripetibili, come l'aumento dei consumi interni, stante la disponibilità di maggior reddito degli italiani, grazie anche ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego e dei metalmeccanici. Quindi l'attenuazione del trascinamento della domanda mondiale, della domanda dei consumi interni e della impermeabilità del mercato interno tedesco, ci rende consapevoli come ulteriori politiche restrittive, legate ad un risanamento cieco, possano deprimere ulteriormente la nostra economia, proprio mentre sta agganciandosi alla ripresa internazionale. Prefigurare per il 2007 un indebitamento netto al 2,8

significa fare una politica da grande coalizione, come hanno indicato gli amici Follini, Tremonti e Berlusconi e non una politica di piccola coalizione, come a giorni alterni indicano Mastella, Ferrero, Di Pietro e quanti altri stanno stanno con un piede dentro e uno fuori da questo Governo. Con una finanziaria 2007, preannunciata con una manovra di 35 miliardi di euro: 20 da destinare al risanamento e 15 alla crescita, di cui 10 miliardi di euro di presumibili entrate e 10 di presumibili tagli, è difficile pensare che questo Governo possa unire l'Italia e concertare con le parti sociali un suicidio politico ed elettorale. Sicuramente prevarranno le vendette sociali, così come è stato per

del sostegno alla ricerca, degli ammortizzatori sociali che avrebbero dovuto correggere la legge Biagi. Alla Confindustria e agli altri elettori italiani, ai quali avete fatto credere ai quali avete fatto credere che il taglio al cuneo fiscale fosse integrale, 5 punti nei primi 100 giorni, costa dieci miliardi di euro. Poi avete ritrattato. I tavoli tecnici stanno studiando interventi selettivi che favoriscano la trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, per non parlare dell'internazionalizzazione delle imprese, della ricerca, del Mezzogiorno e via discorrendo. Comunque andranno le cose, il finanziamento del cuneo fiscale richiede coperture certe ed immediate. Il recupero di entrate, dettate dalla virtuosità dell'intervento, hanno invece un arco di tempo ben superiore all'esercizio finanziario di riferimento.

con tagli alla spesa pubblica, sia con l'aumento dell'IVA, le ricadute negative sui consumi interni che hanno tirato la crescita del 2006, saranno certe e preoccupanti. La vostra strategia deprimerà la nostra economia, altro che crescita.

lavoratore. La logica «più profitti meno salari reali», secondo i teorici della sinistra liberale, dovrebbe trasformarsi in quella «più investimenti e meno consumi». Sindacati, sinistra e Confindustria dovrebbero concertare questo patto leonino. Signor Presidente, gli italiani stanno cominciando a preoccuparsi di Prodi e del suo Governo. Noi siamo preoccupati del fatto che ancora non siamo pronti a soluzioni alternative.

Signor Presidente, questo primo Documento di programmazione economico-finanziaria della nuova legislatura rappresenta una importante novità, non solo per i segnali di ripresa che in esso vengono tratteggiati, ma soprattutto perché questo Documento torna ad avere il ruolo strategico che merita, caratterizzandosi per linearità e chiarezza. L'Italia ha bisogno di passare dalla finanza creativa ad una politica economica seria. C'è un forte bisogno di riprendere fiducia in se stessi. La discussione sul Documento di programmazione economico-finanziaria, che si è sviluppata nel Paese e che ha trovato ascolto nel dibattito parlamentare, ha prodotto una risoluzione che soddisfa largamente le aspettative e risponde alle domande che anche il nostro partito aveva sollevato. Certo su alcuni temi bisognerà produrre un approfondimento in sede di discussione sulla legge finanziaria. La strategia complessiva per il 2007-2011 è costruita intorno a tre pilastri indispensabili: crescita, risanamento ed equità sociale. Nessuno dei tre obiettivi è meno importante degli altri. Il Governo e la maggioranza hanno l'ambizione di realizzare compiutamente i tre obiettivi, così come è scritto nel programma con cui l'Unione si è presentata agli elettori. Nel DPEF si evidenziano i problemi strutturali dell'economia italiana, a cominciare dalla perdita di produttività, soprattutto nell'industria. Il dato è davvero impressionante: mentre nel 1995 la produttività oraria del nostro Paese era del 4 per cento superiore a quella dell'area dell'euro, nel 2005 è inferiore del 3 per cento. In questi dieci anni, il tasso di crescita della produttività in Italia è pari a meno di un quarto di quello europeo. E le cause vanno ricercate nella dimensione media delle nostre aziende, nella scarsa propensione agli investimenti in ricerca e innovazione, nella mancanza di specializzazione in settori tradizionali, come quello manifatturiero, che producono ed esportano beni a basso contenuto tecnologico. Basti pensare che, nella ricerca, la spesa privata in rapporto al PIL è tra le più basse tra i Paesi industrializzati. Di qui la perdita di competitività dell'economia italiana e la perdita di quote di mercato internazionale, tendenza che si conferma per l'anno in corso. Anche quando l'Europa e gli Stati Uniti crescono, noi arranchiamo, scontando così l'allargamento del divario dai Paesi più avanzati. Nel DPEF si prende atto di quanto è accaduto nel corso dei decenni, e se ne conclude che bisogna intervenire sui fattori che determinano la crescita. È un compito che spetta alla parte pubblica: il mercato non è autosufficiente, non lo è mai stato. Il mercato, lasciato a se stesso, produce distorsioni e disparità economiche, ma anche intollerabili squilibri sociali. Questo Governo e questa maggioranza hanno anche il dovere di ricostruire, un po' per volta, quel senso di appartenenza, quell'*idem sentire* che né le leggi *ad personam* né i condoni sono riusciti ad erodere del tutto. È questo il grande insegnamento che ci consegna il *referendum* costituzionale, di cui dobbiamo far tesoro nelle scelte programmatiche come nei provvedimenti quotidiani. Ereditiamo una finanza pubblica disastrata, per sanare la quale ci siamo impegnati davanti alle istituzioni europee e agli organismi internazionali. A tal proposito, si potrebbe facilmente notare come queste istituzioni ed organismi abbiano taciuto di fronte alle evidenti bizzarrie del precedente Governo, o che comunque siano state fin troppo accondiscendenti. Ora si chiede a noi di porre rimedio, immediatamente, ai danni che si sono prodotti in cinque anni di Governo Berlusconi e che, purtroppo, dispiegheranno i propri pesanti effetti ancora a lungo. È una ben strana disparità di trattamento, e pur nella consapevolezza della necessità di intervenire con misure rigorose e credibili, crediamo che non bisogna lasciarsi ingabbiare dalle eccessive rigidità dei parametri di Maastricht. Il pericolo reale è che si rischi di uccidere la ripresa prima che essa si sia affermata: non possiamo permettercelo. Non lo sopporterebbe l'economia, non lo reggerebbero i cittadini, i lavoratori, i pensionati, i disoccupati, l'estesa platea dei precari. Ed è per questo motivo che riteniamo che l'azione di risanamento possa dispiegarsi in un arco temporale più largo tale da consentire che il risanamento avanzi di pari passo con le azioni di sviluppo e nel rispetto dei criteri di equità e di giustizia sociale. Positivo mi pare altresì l'accento posto sulla lotta all'evasione e all'elusione fiscale, i cui proventi saranno destinati al sostegno allo sviluppo e per le infrastrutture, quelle utili al Paese, abbandonando definitivamente quelle inutili e dannose come il Ponte sullo Stretto. È il segno di una inversione di tendenza rispetto al recente passato contraddistinto dalla logica dei condoni di ogni genere che hanno ridotto significativamente le entrate del nostro Paese. Bisogna continuare su questa strada, segnare la discontinuità rispetto a quel «pensiero unico» che sembrava fino a qualche anno fa aver definitivamente vinto. In tal senso, giudichiamo positivamente le indicazioni che il DPEF trae dall'analisi dei dati sulla composizione della disoccupazione, da cui deriva la scelta di favorire la crescita occupazionale attraverso interventi per il miglioramento quantitativo e qualitativo del lavoro femminile, che insieme a quello giovanile rappresentano i pilastri per il rilancio complessivo del nostro Paese. Ci sono punti di particolare delicatezza, in quanto capaci di aprire la strada ad esiti tra di loro contraddittori, come ha sottolineato il ministro Ferrero in Consiglio dei ministri. Penso, ad esempio, alla spesa pensionistica e, dall'analisi del DPEF, non si evidenzia a nostro avviso la necessità di mettere mano ad una riduzione della spesa previdenziale, soprattutto dopo gli interventi del 1992 (riforma Amato) e del 1995 (riforma Dini), e soprattutto in considerazione

Alcuni dati negativi sul rapporto tra spesa pensionistica e PIL evidenziano come nel nostro Paese, a differenza di tutti quelli più avanzati, sulla previdenza incidono voci che invece dovrebbero essere a carico dell'assistenza e, quindi, della fiscalità generale. Una separazione tra previdenza ed assistenza viene segnalata come esigenza nella risoluzione dell'Unione che ci apprestiamo a votare. L'innalzamento obbligatorio dell'età pensionabile è assolutamente antitetico alla costituzione di uno Stato sociale moderno ed efficace, capace cioè di incidere veramente sulle cause di disparità sociali e di dare attuazione all'articolo 3 della Costituzione. Già da questa discussione, insomma, occorre aprire il tema della ridefinizione strutturale del *welfare State*, che deve essere visto e pensato come costruttore di ricchezza economica, oltre che sociale, sul modello delle più avanzate democrazie europee. Invece, negli ultimi anni, il fondo per le politiche sociali è stato ripetutamente tagliato, come se la spesa sociale del nostro Paese non fosse già inferiore alla media dei paesi dell'Unione Europea. Bisogna altresì intervenire sul tema della distribuzione del reddito, in Italia, negli ultimi anni, ha visto crescere le disuguaglianze. Negli ultimi quattro anni la ricchezza si è spostata verso le classi di reddito più alte: uno sbilanciamento in favore del lavoro autonomo e a detrimento dei redditi delle famiglie composte da operai ed impiegati. Le famiglie più ricche hanno avuto un incremento dei redditi reali pari a circa 9.000 euro all'anno, mentre la perdita per le famiglie di lavoratori dipendenti è stata di oltre 1.400 euro. Se si tiene conto dell'incidenza percentuale di questi numeri su redditi molto diversificati tra loro, ci si rende conto della sofferenza profonda in cui sono costrette le famiglie meno abbienti del nostro Paese. Bisogna che il Governo e la maggioranza assumano questo dato prioritario. Dobbiamo inoltre impegnarci a definire compiutamente i livelli essenziali delle prestazioni sociali, che vanno accordate con i livelli essenziali di assistenza sanitaria, integrando opportunamente politiche sociali, sanitarie, formative e del lavoro, che costituiscono, insieme alle politiche tariffarie e della casa, la condizione indispensabile per l'inclusione sociale. Si deve aprire una riflessione sulla sperimentazione del reddito minimo di inserimento inopinatamente chiusa dal Governo Berlusconi; basti pensare che l'Italia e la Grecia sono i soli due paesi dell'Unione Europea tuttora privi di una misura di contrasto alla povertà di carattere universalistico, nonostante le indicazioni europee insistano da sempre sul punto. La cartografia sociale del Paese si sovrappone a quella territoriale. La questione del Mezzogiorno è sempre aperta ed è sempre più grave, poiché la distanza dal resto del Paese e dall'Europa è ulteriormente aumentata. I dati dell'ultimo rapporto SVIMEZ presentano tutti gli indicatori di crescita negativi nel Mezzogiorno e finalmente, dopo anni di silenzio, il Governo dell'Unione traccia le linee di un intervento organico per il rilancio dell'economia meridionale, che privilegia le misure a sostegno delle aziende che innovano e producono «lavoro buono». Nella risoluzione si fa esplicito riferimento alla valorizzazione delle risorse umane, della ricerca e dell'innovazione, nonché alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali: un Mezzogiorno che abbandona la logica della rincorsa del costo del lavoro al prezzo più basso e che diventa grande laboratorio aperto ad un Mediterraneo di pace. Grande attenzione riceve la questione ambientale, che non può essere scissa dai temi dello sviluppo; i primi passi del Governo sono stati incoraggianti. L'attuazione del Protocollo di Kyoto, il sostegno effettivo alle fonti rinnovabili, la valorizzazione dei beni comuni, l'affermazione della valutazione ambientale strategica, l'introduzione di indicatori ambientali, che affiancheranno quelli macroeconomici, e l'adozione di un sistema di contabilità ambientale rappresentano una vera inversione rispetto alle politiche ambientali fin qui condotte.

lo *status* di diritto fondamentale. Stiamo già intervenendo per sterilizzare gli effetti del cosiddetto codice ambientale. La discussione fin qui svolta ha spostato in avanti il dibattito rispetto al momento dell'approvazione del DPEF nel Consiglio dei ministri. Molto è stato fatto, altro ci attendiamo dalla legge finanziaria, ma già nella risoluzione si colgono gli elementi correttivi rispetto ad una lettura troppa rigida del risanamento. Il Gruppo Rifondazione Comunista-Sinistra Europea

*(AN)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ovviamente dobbiamo esprimere un voto sul testo scritto del Documento di programmazione economico-finanziaria che ci è stato sottoposto, e non sulle pie intenzioni che da qualche parte qualche esponente più saggio di questa maggioranza ha tentato di contrabbandare in quest'Aula. Ciò che ci è parso chiaro è che questo Documento di programmazione economico-finanziaria, che parte come un documento da centro studi, in realtà sottintende un preciso patto politico con il blocco sociale. È vero, amici della maggioranza, non c'è la politica dei due tempi; infatti, c'è la politica di un tempo solo. E quel tridente, che è crescita, risanamento finanziario...

più volte fuori e dentro quest'Aula - crescita, risanamento, equità sociale - viene smascherato; la crescita non c'è, l'equità sociale non c'è. Resta un mero risanamento finanziario, senza sviluppo, senza occupazione, senza equità sociale; per di più, con una *overdose* di equilibrio finanziario, perché si pone come obiettivo programmatico non il sacrosanto contenimento del *deficit* al di sotto del tre per cento, ma addirittura il suo azzeramento; non la stabilizzazione del rapporto debito pubblico-PIL ma la riduzione rapida al di sotto del 100 Questi due obiettivi di risanamento finanziario sarebbero chiaramente accettabili e da perseguire se le contropartita non fosse la crescita asfittica, la disoccupazione che non scende e addirittura controbilanciata con un obiettivo di inflazione che nella media europea è del 2 per cento e nel DPEF viene posto all'1,5 per cento. Vogliamo essere eccessivi sul lato del risanamento finanziario ma dimentichiamo che sarebbe un risanamento finanziario fragile e precario perché senza la crescita neanche quel risanamento finanziario è possibile.

di sostegno alle famiglie, a reddito medio-basso e alle famiglie numerose - come sapete, noi sosteniamo il quoziente familiare in tema di piccole e medie imprese. È palese lo scambio dei cinque punti di riduzione del cuneo - non si sa bene se sia fiscale o contributivo che per tre quarti va a grandi imprese, grandi banche e grandi assicurazioni e si fa silenzio sulla riduzione dell'IRAP alle piccole e medie imprese. Ancora, per il silenzio sul Sud; Sud; è francamente paradossale che la maggioranza si sia vista costretta a presentare in quest'Aula l'emendamento 2.1, che dimostra palesemente quale sia la carenza nel DPEF dei temi sul Mezzogiorno, al punto tale che le maggioranza ha introdotto questa sera, all'ultimo momento, un emendamento che avrebbe in qualche misura pur se con alcuni aspetti criticabili - rafforzato le linee sul Sud; un emendamento che non è riuscita neanche a far approvare. E in cambio di tutto questo cosa riceviamo? L'introduzione ieri di uno Stato che fa da Grande fratello, della tracciabilità del cittadino, e questa notte, mentre nel DPEF si annuncia sostegno all'istruzione, alla ricerca, all'università, questa notte voi della maggioranza, voi del Governo, nel decreto Visco-Bersani avete tagliato i fondi all'istruzione, all'educazione, e alla ricerca. Lo ha detto ieri il collega Valditara in quest'Aula, e gli avete dato del bugiardo. Oggi il Presidente della Conferenza dei rettori pubblicamente denuncia: i tagli passati questa notte nel primo atto di politica economica di questo Governo. Allora, il buonismo e le pie intenzioni, smentite dai fatti concreti, ovviamente ci portano ad esprimere un voto negativo a questo decreto.

Ho la sensazione che se questo DPEF per voi non è il libro dei sogni, la finanziaria a settembre per voi diventerà il libro degli incubi. Allora, mentre il vostro ministro Ferrero non ha votato questo DPEF, mi chiederò come potrete votare a settembre una finanziaria che annuncia 35 miliardi di tagli su sanità, pensioni, pubblico impiego ed Enti locali. Ovviamente, questo è un problema interno alla vostra maggioranza. Da parte nostra saremo sempre attenti alle sorti del Paese e a quelle difficili decisioni di politica economica che debbono combinare risanamento finanziario, sviluppo, riequilibrio territoriale, sostegno al Sud, ma non siamo disposti a farci prendere in giro dai titoli di un libro privo di contenuti, anzi con contenuti contraddittori rispetto agli stessi titoli, come il decreto che avete approvato voi questa notte dimostra nel caso specifico - e non solo - delle spese per istruzione, ricerca e sviluppo. Convintamente esprimo il voto

dichiaro a nome del Gruppo Forza Italia il voto favorevole alla risoluzione n. 1. che, a suo avviso, tutti sarebbero d'accordo, quanto meno, sull'entità finanziaria complessiva della manovra che è lumeggiata nel DPEF: strana affermazione, signor Presidente, dato che da quanto risulta agli atti, nemmeno la maggioranza e nemmeno il Governo è d'accordo con sé stesso.

che verranno effettivamente adottate». Questo vuol dire che il Governo non sa oggi che tipo di misure verranno prese. *(Applausi dai Gruppi FI e AN).* Forse sta cercando di ripetere quello che è stato fatto nel 1996, quando l'allora Presidente del Consiglio Prodi voleva fare una manovra più ridotta, poi andò in Spagna da Aznar, tornò con le pive nel sacco e fu costretto a cambiare la manovra in corso d'anno. Forse è un *déjà vu* che continuerete a dare al Paese, il Governo stesso non sa che cosa effettivamente vuole, non vedo perché ci si dovrebbe mettere d'accordo sulla quantità della manovra. In realtà, la manovra così come è descritta nel DPEF è di entità assolutamente esagerata esagerata ed inadeguata e deriva da alcune *expertise* fatte, non come si dovrebbe usare da organismi di ricerca come l'ISTAT, la Corte dei conti o la Banca d'Italia, ma da ma da un seppur bravissimo professore di nomina governativa, che si è limitato a comportarsi come farebbe qualunque oste a cui si chiede della bontà del vino che vende. del vino che vende. Questa manovra, chiaramente esagerata nelle sue quantità, non ha altro scopo se non quello di lasciare al Governo le mani libere per fare qualunque cosa nei prossimi mesi e per cercare di modificare l'andamento dell'economia italiana e della sua finanza pubblica. Tra l'altro, essa ha un contenuto intimamente contraddittorio, perché, se è vero quello che dice il Governo di volere mirare all'equità, allo sviluppo e al risanamento economico, sicuramente uno di questi obiettivi è mancante, perché la manovra che ha caratteristiche assolutamente recessive: 35 miliardi di euro, circa 70.000 miliardi di vecchie lire, sono una cifra imponente, rappresentano la seconda manovra dopo quella di Amato del 1992. Una manovra con simili caratteristiche recessive ha l'effetto - e lo dice lo stesso DPEF - di comportare un tasso di sviluppo per il 2007 inferiore a quello che sarebbe stato in assenza di manovra. Quindi, quando il Governo mette le mani sulla finanza pubblica produce danni all'economia, se non sa dove mettere le mani e se si comporta come un elefante nelle cristallerie. Ma la domanda principale - l'ha detto anche poc'anzi il rappresentante del Governo - è quella se il Governo, dopo aver enunciato una manovra di tale rilievo sarà in grado di realizzarla. Il Governo dichiara di voler intervenire nei principali settori di spesa: è in grado di farlo? Parla di pensioni, ma già il Ministro dell'economia ha detto che l'innalzamento dell'età pensionabile potrà avvenire solo su base volontaria, cioè non avverrà mai, e il collega di Rifondazione poco fa ha detto che le pensioni non si toccano. Il Governo parla di intervenire sulla questione degli enti locali, ma già nel DPEF dice che si vuole passare da un sistema di limitazione della spesa, ad un sistema di saldi, cioè in sostanza vuole dare mano libera agli enti locali per aumentare le tasse, che saranno ancora una volta pagate dai cittadini! *(Applausi dal Gruppo* *FI).* Il Governo dice che bisogna intervenire nel settore della spesa sanitaria, ma prontamente il Ministro della salute che occorre introdurre i *ticket* sui ricoveri per i più abbienti, cioè ancora una volta non si vuole regolamentare la spesa, ma si vuole aumentare la tassazione a danno dei ceti medi.

tacciono, come stanno facendo su tutto ciò che avviene e che viene determinato da questo Governo. *(Applausi dal Gruppo FI)*. In sostanza, signor Presidente, se guardiamo al lato del contenimento della spesa, già adesso - siamo a luglio e dovremo attendere settembre - la manovra si va sfarinando in mano al Governo: ciò che resta, ahimè, è esclusivamente l'aumento delle tasse e della pressione fiscale. Non lo dico dal punto di vista della opposizione, ma lo dico leggendo la risoluzione di maggioranza sul DPEF, la risoluzione di maggioranza sul DPEF, la quale unisce una serie di spese *a gogò, à la carte*, con alcune impostazioni esclusivamente basate sull'aumento delle tasse. Certo, c'è il solito ricorso alla lotta all'evasione, ma c'è anche la tassazione delle rendite finanziarie: lo avevamo detto in campagna elettorale e adesso lo vediamo scritto. una piccola domanda: quale Governo irresponsabile al mondo va dichiarando, cinque mesi prima di realizzarlo, che aumenterà la tassazione sulle rendite finanziarie, con l'unico effetto di far scappare i capitali? *(Applausi

che significa che vorrà aumentare la tassazione sui ceti medi, su coloro che lavorano e producono. E poi afferma, simpatica espressione, che si tasseranno le attività speculative e meno quelle produttive: ma cosa è speculazione e cosa produzione? Quel che fanno gli altri è speculazione, per caso? E poi, l'abbiamo visto nel decreto-legge n. 223 del 2006, la realtà è quella di costituire un meccanismo di conoscenza talmente pervasiva delle posizioni fiscali e patrimoniali di ciascun contribuente italiano, in una sorta di Grande fratello, per precostituire la base per arrivare un domani ad una tassazione patrimoniale dei patrimoni di ciascun cittadino italiano, il che, ovviamente, è assolutamente inaccettabile. La questione, come si è detto, è chi sarà in grado di votare una manovra di questo genere, chi sarà in grado di sostenerla: il Governo, in realtà, oggi non è in grado di saperlo. proposito, basta leggere la risoluzione di maggioranza, perché essa (ed è la prima volta che accade una cosa del genere) precisa già a luglio che si invita il Governo a presentare una nota di aggiornamento del DPEF a settembre, con le integrazioni al quadro degli elementi di ordine quantitativo concernenti in particolare l'entità e la composizione della manovra da realizzare per il 2007. Ciò vuol dire che, al 26 luglio, il Governo non sa cosa fare e si riserva ancora una volta le mani libere a settembre per vedere che cosa sarà riuscito a fare nel frattempo e se avrà o meno una maggioranza. Cari signori del Governo, dalla lettura di queste carte, dagli atti, una cosa è chiara: o il Governo non sarà in grado di realizzare la manovra che ha illustrato con con qualche riserva adesso, a luglio, nel Documento di programmazione o non potrà far altro che seguire la strada che ha già percorso con il decreto-legge n. 223 del 2006, aumentare la pressione fiscale. D'altronde, è connaturale ad un Governo che debba in qualche modo mantenere un sistema di potere - che fino adesso gli ha garantito appunto il potere - il succhiare sempre più risorse ai contribuenti per destinarle a chi lo sostiene. L'esempio del decreto-legge n. 223, che, sostanzialmente, con la scusa delle liberalizzazioni, tende a finanziare in modo molto corposo il mondo delle cooperative ne è la prova provata. Il vice ministro dell'economia, l'onorevole Visco, ha detto che il Governo realizzerà il suo programma e che non ha bisogno di nessuno: la maggioranza comanda e la maggioranza andrà avanti. Buon lavoro, onorevole Visco, buon lavoro al Governo. Proceda pure il Governo in splendida solitudine, senza ascoltare il Paese che lavora, senza ascoltare il Paese che produce, senza ascoltare il Paese che risparmia, senza ascoltare il Paese che investe, senza ascoltare il Paese che aspira a maggiore libertà, anche economica, e che spera in un domani migliore. Proceda pure il Governo, sordo e cieco verso il suo destino.

che tiene insieme il documento, la sua discontinuità con le politiche precedenti e l'orizzonte che lo giustifica come documento di legislatura che dovrà sostenere l'azione di Governo per cinque anni. Questo è il senso del DPEF, che ne giustifica la funzione, finché la si riterrà utile. Si tratta di un impianto coerente, con orientamenti definiti di politica pubblica, nient'affatto generici, né minimalisti, anzi molto ambiziosi (a dire il vero siamo stati accusati di tutto, di essere evanescenti, minimalisti, esagerati). Proprio per questo è difficile da realizzare per la sua complessità e la sua ambizione, ma i fatti dimostreranno che l'obiettivo è raggiungibile. Un obiettivo ambizioso è essenziale per far uscire il Paese da una crisi economica grave e da una sofferenza sociale altrettanto grave, per farlo ripartire, come si dice, per rimettersi al passo, solo con qualche enfasi, purtroppo. La gravità della situazione che abbiamo ereditato richiede misure coraggiose e il DPEF le propone precisamente, anche se con un carattere di quadro proprio del documento, sulle tre direzioni qui più volte ricordate: risanamento, sviluppo ed equità.

linee si potranno raggiungere gli obiettivi e troveranno senso anche gli specifici provvedimenti. Credo che questo sia messaggio debba essere spiegato e interiorizzato da tutti, nelle nostre politiche e nelle azioni degli operatori. qualche esempio molto semplice e chiaro sui tre punti. Anzitutto, la ripresa della crescita; questa è una priorità, checché ne pensino le opposizioni, con argomenti a dire il vero inconsistenti. Solo la crescita permette di generare le risorse necessarie per risanare i conti pubblici e per aumentare il benessere personale e sociale. Può sembrare un'affermazione ovvia ma non lo è affatto, è un'affermazione importante che si traduce in orientamenti precisi. Questi orientamenti segnano una netta inversione di tendenza rispetto alle politiche della scorsa legislatura, che erano fondate su diagnosi e previsioni poco credibili e su una politica di sostegno alla domanda di riduzione fiscale di dubbia credibilità e infatti non realizzata, con risultati fallimentari che sono sotto gli occhi di tutti. La politica economica del DPEF, invece, si incentra sul lato dell'offerta e punta a correggere i fattori di debolezza del nostro sistema economico, tutti i fattori che hanno questa debolezza. L'intervento più immediato, quello che si vede immediatamente è l'intervento sul costo del lavoro che ha dimensioni senza paragoni nel passato e che serve sia a dare una scossa alle imprese, che un sostegno ai redditi dei lavoratori. Ma questo provvedimento non va visto solo come una riduzione del costo del lavoro,

sull'innovazione che possiamo e dobbiamo puntare, come si dice nel DPEF. Questa indicazione ha già trovato un'attuazione nelle misure approvate con il decreto Bersani-Visco

avremmo un atteggiamento punitivo nei confronti dei ceti produttivi. Non solo lungi dall'avere questi intenti, in realtà la linea che proponiamo nel DPEF, e che coerentemente porteremo avanti nei prossimi anni, è anni, è prioritariamente quella di sostenere gli attori e i fattori della produzione, le imprese per la loro competitività e il lavoro, con una occupazione di qualità.

non per motivi di carattere spicciolo-rivendicativo posti in contrapposizione al Nord o alla sua presupposta questione, ma per la ragione fondamentale che un rafforzamento di interventi in questa direzione, trascurati invece in questi anni, è essenziale per la crescita dell'intero Paese. Questa è la linea indicata già nel programma di Governo del centro-sinistra che noi vogliamo sviluppare. Poi le misure appropriate per raggiungere raggiungere questo risultato - che possono e devono riguardare l'aumento e la qualificazione degli investimenti fino alla fiscalità di vantaggio - andranno individuate e rafforzate nella sede propria, e cioè nella legge finanziaria. Le politiche di crescita indicate nel Documento non propongono uno sviluppo qualsiasi, ma uno sviluppo caratterizzato da alta qualità tecnica e alta qualità sociale. Questo sottolinea il nesso tra le due linee d'intervento cui accennavo all'inizio del mio intervento: alta qualità tecnica, perché appunto non possiamo competere sulla riduzione dei costi ma sull'innovazione, sulle risorse umane e quindi sul loro potenziamento attraverso politiche all'altezza degli obiettivi della società della conoscenza; qualità sociale, che si estrinseca nelle varie misure di politica pubblica e, in particolare, nelle politiche pubbliche di carattere sociale. Anche in questo caso la connessione tra la linea dello sviluppo e la linea dell'equità non è declamata, ma si vede in misure concrete che ovviamente sono impegnative ma che sono indicate in modo coerente, a cominciare dalla scelta di utilizzare la riduzione del costo del lavoro per aumentare la buona occupazione, cioè l'occupazione stabile, l'attenzione sulle misure che mirano a costruire un *Welfare* non solo universalistico ma attivo, capace di rafforzare la coesione sociale - un'altra parola chiave del nostro messaggio che è sconosciuta, purtroppo, alla nostra opposizione - con la coesione sociale e la fiducia nel futuro. Si tratta di interventi che toccano punti impegnativi, come la riforma degli ammortizzatori sociali, essenziali sia per il sostegno ai diritti delle persone, ma anche per rendere praticabile una mobilità essenziale in un sistema produttivo e sociale in grande mutamento.

di un obiettivo essenziale, come sappiamo, perché il successo del risanamento è una condizione della crescita: non si danno Paesi che crescono che sani da questo punto di vista. Per altro verso voglio sottolineare che l'efficacia e la stabilità del risanamento sono infine affidate alla capacità del sistema di reagire alla crisi e riprendere la via del sviluppo.

sia sulla qualificazione e sul contenimento della spesa. Dal primo punto di vista - è stato detto, ma lo sottolineo - si punta su un regime di tassazione più giusto, ripulito dai mali dell'evasione e dell'elusione, mali sociali ed economici. sociali ed economici. Il DPEF non si nasconde che la gravità degli squilibri finanziari rende necessari interventi sulle strutture portanti della spesa pubblica (i quattro comparti indicati), ma segnala la possibilità e la necessità che questi interventi non impoveriscano l'essenziale funzione di solidarietà in questi settori di promozione delle crescita, di forniture di beni pubblici La nostra bussola è intervenire per correggere le inefficienze, le arretratezze, le duplicazioni e le sovrapposizione di funzioni, legate a un malinteso decentramento, e - ebbene sì - ai costi della politica:

La coerenza, poi, si verificherà nell'azione di Governo, giorno per giorno, nel periodo della legislatura che è l'orizzonte del DPEF e della nostra maggioranza. Siamo convinti che questo disegno ci sosterrà

per l'elezione del Consiglio d'Europa e dell'UEO. È una votazione sola, quindi se la faremo con serenità e tranquillità finiremo in un attimo. Procediamo

in modo che i segretari possano verificare le postazioni. Bisogna cercare di evitare di coprire le tessere con gli oggetti più disparati.

**Votazione a scrutinio segreto per l'elezione dei membri effettivi e supplenti della delegazione italiana all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e dell'Unione L'ordine del giorno reca la votazione per l'elezione dei membri effettivi e supplenti della delegazione italiana all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e dell'UEO. Tale votazione avverrà, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento, a scrutinio segreto sulle seguenti liste di candidati formate su designazione dei Gruppi parlamentari. Membri effettivi, senatori: Boccia Maria Luisa, Cantoni, Dell'Utri, Formisano, Manzella, Pinzger, Silvestri, Soliani e Valentino. Membri supplenti, senatori: Barbato, Del Roio, Livi Bacci, Malan, Mele, Morselli, Nessa, Pellegatta e Sinisi. I senatori favorevoli alle liste proposte voteranno sì. I senatori contrari voteranno no. I senatori che intendono astenersi si comporteranno di conseguenza.